in cui i vantaggi vanno sempre più ai privati ed il bene pubblico è sempre meno nelle mani del pubblico; è fondata sul lavoro, un lavoro che già era in crisi e che con gli ultimi provvedimenti, approvati in questa legislatura, è stato ulteriormente massacrato come valore e non solo come entità e come quantità;

Questa sovranità effettivamente appartiene più ai colleghi che al popolo e apparterrà sempre meno al popolo, perché con questo disegno di legge elettorale vengono fissate delle regole d'ingaggio.

quando noi siamo entrati in Senato, siamo entrati con una legge che già nel nome indicava la dignità con cui entravamo, una legge con cui non siamo stati scelti e che che è stata dichiarata incostituzionale. Credo che tutti abbiamo sofferto, o almeno io ho sofferto per il fatto di non essere stata scelta e di non poter avere un'idea chiara e concreta di quante persone affidavano a me personalmente il compito di rappresentarle.

e se gli fa schifo il fatto di non poter votare in modo chiaro e trasparente e indicare chi vuole che lo rappresenti, può sempre rimanere a casa sua. Questo è il punto centrale:

pensiamo a quello che serve al Paese. Questa è veramente l'evocazione di una scena surreale, perché in realtà quando decidiamo, ovvero quando decidono di votare un emendamento, lo fanno perché hanno qualcuno che dà loro un'indicazione. Il bene del Paese è veramente l'ultima delle preoccupazioni. Personalmente quando voto un emendamento cerco di capire cosa c'è scritto. Vedo che gli altri invece votano secondo indicazioni di partito. L'unico che ho visto cambiare idea è stato il ministro Orlando in Commissione (questo gli va riconosciuto),

i partiti, tutti i partiti, formulano regole d'ingaggio che sono modellate su di loro e non sugli elettori, perché nel momento in cui viene eliminata la preferenza, nel momento in cui vengono attivati meccanismi di ricasco dei voti in modo surrettizio e truffaldino, è chiaro che si inganna l'elettore. Così l'elettore è libero di non andare a votare e infatti non ci va. Ma questo ai partiti non interessa; anzi, è meglio, perché la partecipazione è qualcosa di difficilmente controllabile. Non gliene può fregare di meno se non partecipano. Il fatto che i cittadini stiano a casa non è rilevante; anzi, meno vanno a votare più sono controllabili, perché sono quelli che indirettamente o direttamente sono a libro paga,

La faccenda delle preferenze non riguarda solo l'elettore in modo diretto e quindi la possibilità di scegliere. La faccenda delle preferenze è qualcosa che riguarda ancora di più l'eletto,

Quindi, le preferenze servono ancora di più per modellare il comportamento dell'eletto che non per dare all'elettore l'immediata libertà di scegliere. Così cadono tutti gli argomenti con cui non si vogliono concedere le preferenze, nella misura in cui sono sostenuti da una sostanziale sfiducia nei confronti del popolo e rivelano un sostanziale disamore, anzi un fastidio per tutti i meccanismi democratici. Questa sovranità deve infatti essere gestita essere gestita come un patrimonio personale, perché chi è qui dentro aspira a ritornarci, a rimanerci e a esercitare del potere, perché in ben poche persone qui dentro ho visto quell'umiltà e quel rispetto per l'elettorato che è invece l'unico che può animare un amore vero per la democrazia. Il termine della governabilità è ridicolo e grida vendetta, perché la governabilità è strettamente collegata alla percezione di fare il bene del Paese. Mi si dirà che i partiti presentano dei programmi. Al di là del fatto che non ho ancora visto nessuno qua dentro rispettare un programma, qui non c'è neanche rispetto dei principi. Faccio un esempio: sono un elettore che crede nella scuola crede nella scuola come il polmone della crescita e dello sviluppo dei singoli cittadini e del Paese. Quindi legittimamente penso che, al di là dei programmi,

peggiora le condizioni della legge Gelmini, ma che contraddice anche dei principi solidissimi. Non si tratta, quindi, solo di programma, ma anche di principi. Ho fatto questo esempio, ma avrei potuto farne tanti altri. Cosa deve Cosa deve fare un elettore a questo punto? Di chi si deve fidare? Per quale ragione l'elettore dovrebbe essere meno capace di scegliere i suoi rappresentanti di quei segretari di partito, di quei potentati che sono all'interno dei partiti o dei movimenti

Per quale motivo? Dov'è la ragione per cui il soggetto che appartiene al popolo dovrebbe rinunciare a scegliere? Qui dentro chi ha dimostrato di essere più capace di scegliere? Questo è il segno della mancanza di ciò che servirebbe di più per poter stare qui dentro, cioè un amore autentico per le prime righe della Costituzione. se la sovranità appartiene al popolo, ciascuno agisce in nome e per conto del popolo, non in nome e per conto di sé stesso, della propria struttura di partito o di movimento e per la sopravvivenza della propria visibilità e del proprio potere. Tutto questo naturalmente non c'è nel disegno di legge in discussione. Ancora una volta viene persa un'occasione, ma non si poteva neanche immaginare che potesse essere colta. Purtroppo i cittadini confondono le persone che interpretano le istituzioni con le istituzioni stesse. Purtroppo, perché i cittadini dovrebbero essere i primi a fare questa distinzione. È un po' comportarsi come Gesù nel tempio: prendere in mano la frusta e sbattere fuori dalle istituzioni coloro che non ne sono degni. Invece saranno costretti ad accettare una legge che,

per motivi forse simili e forse diversi; non ne sarò complice anche con rammarico, pensando che purtroppo il popolo non sembra molto intenzionato a riprendersi le istituzioni. Purtroppo, quella grande spinta alla partecipazione che mi aveva portato qui

Bisogna ricominciare tutto da capo, forse dalla scuola, forse dai giovani, l'unica fetta di popolo che in quest'Aula non è mai stata nominata con rispetto. Forse bisogna cominciare dalle persone che stanno peggio, forse bisogna ricominciare proprio fuori da queste Aule.

Rispetto al sistema attualmente in vigore, ossia l'Italicum alla Camera e il Porcellum al Senato, debitamente rimaneggiati dalle sentenze della Corte costituzionale, questa nuova proposta riapre la porta alle coalizioni, quindi danneggia quelle forze politiche non coalizzabili (per volontà propria o altrui) come il Movimento 5 Stelle, che infatti ha già bollato questa proposta come incostituzionale, rifiutandosi anche solo di prenderla in considerazione. Non danneggia i piccoli partiti, in teoria: anzi, alla Camera consente loro di riagganciare un partito più grande in una coalizione, magari contrattando delle candidature nei collegi uninominali (come avveniva con il Mattarellum); inoltre rende loro la vita più facile anche al Senato, persino nell'ipotesi in cui restino fuori da qualsiasi coalizione: con la legge attualmente in vigore dovrebbero superare ben l'8 per cento regionale per ottenere seggi. La contrarietà di MDP e di Fratelli d'Italia si può invece spiegare in altro modo: essendo già certi di superare le soglie di sbarramento vigenti, contavano su un sistema per cui ciascun partito si misura da sé con il voto e, dopo le elezioni, può far pesare i suoi consensi; un sistema in cui vi siano (anche solo parzialmente) i collegi uninominali costringe entrambi a un coordinamento pre-elettorale con partiti più grandi, con cui i rapporti potrebbero essere tutt'altro che benevoli (è il caso di MDP nei confronti del PD) oppure col rischio di raccogliere le briciole in una competizione riservata ad altri (ad esempio tra Lega e Forza Italia, a scapito di Fratelli d'Italia). Noi dell'Italia dei Valori, quando lo scorso dicembre il Capo dello Stato ha ritenuto di affidare l'incarico di Presidente del Consiglio a Paolo Gentiloni Silveri, abbiamo assunto l'impegno di mettere in sicurezza il Paese e le nostre comunità. A quel Governo è stato dato, anche grazie al nostro voto, il mandato di condurre il Paese al voto con una legge elettorale costituzionalmente legittima e omogenea per Camera e Senato. Una legge capace di eleggere un Parlamento che sia espressione dell'articolazione plurale e della complessità politica italiana. Una legge in grado di favorire le aggregazioni politiche culturalmente omogenee. L'attuale proposta, approvata con larga maggioranza alla Camera dei deputati e in discussione in Senato, per quanto non sia esattamente quanto noi dell'Italia dei Valori e molti dei presenti in quest'Aula avremmo voluto, è fuori ombra di dubbio una sostituzione efficace del pasticcio normativo delle leggi incostituzionali preesistenti, ampiamente censurate dalle decisioni dell'Alta corte. Non dimentichiamoci che la definizione di collegi uninominali, lo sbarramento ridotto al 3 per cento e la possibilità di formare coalizioni politiche, associate all'armonizzazione dei sistemi elettivi di Camera e Senato, rappresentano indiscutibili passi in avanti. Ho sentito parlare in quest'Aula colleghi che hanno paura che questa legge porterà a un Governo di coalizione che vedrà insieme il PD con Forza Italia e ALA; forse questo potrà essere evitato convincendo gli elettori, soprattutto i tanti indecisi e coloro che non andrebbero a votare, a premiare quelle formazioni politiche, seppure piccole, che si sono messe in coalizione con il solo intento di difendere i valori nei quali credono,

Io per un po' ho mangiato in quel trogolo democratico del Movimento 5 Stelle e per fortuna mi sono solo intossicato e non avvelenato a morte. Egli ha anche aggiunto che il Paese è allo stremo, che saranno votate le persone che saranno disposte ad alzare la mano a bacchetta saremo disposti a entrare in queste Aule con il vestito da burattini. Ecco, vedete, questo spesso è il linguaggio che si legge sul *web*; emerge il linguaggio dell'odio, il ritratto che ne viene fuori è quello di fanatici dediti completamente alle loro idee: un fanatico il cui unico interesse è per una fede, per un'idea; pensa di agire per il bene dell'altro, ma in realtà vuole un mondo in cui non c'è più l'altro. Le strade per uscire da tutto questo sono la buona cultura e la buona politica; in una parola, più Stato di diritto e più cultura. come in molte altre, il problema è che non si analizzano i fatti nella loro complessità, ma secondo uno schema molto semplice: chi è il colpevole, chi dobbiamo mettere alla gogna, su chi dobbiamo scaricare tutte le responsabilità. La caccia del colpevole anche quando non c'è reato è diventata la caccia principale dei *social network*, dove tutto viene vissuto come un processo con condanna annessa: il lancio delle pietre virtuali contro il reo. Oppure quello che ho sentito dire da Crimi che dice che: «si fanno le regole in base ai sondaggi». Forse non si ricorda le regole che cambiano in corso d'opera come alle elezioni della Marika Cassimatis a Genova, seguite dal memorabile commento del professore in filosofia e storia Morra, che ha così commentato la decisione irrevocabile del capo: cogliere, capire razionalmente, ci porta sempre più ad affiancare all'intelligenza razionale una capacità di capire attraverso la fiducia, di "intuire". La mia intuitività mi suggerisce di fidarmi di Beppe, oggi come in tante altre occasioni». In pratica quando gli viene meno la capacità di comprendere razionalmente, si affida con la sua intuitività a Beppe Grillo, il quale da parte sua chiede ai militanti di fidarsi a prescindere.

Il ricambio dei *leader* è rapidissimo e l'imprevedibilità è la caratteristica principale della scena politica internazionale. Tutto questo, per me, non è dovuto né a questa né ad un altro disegno di legge elettorale, ma ad un fatto ben più grave con il quale ci dobbiamo rapportare: l'imprevedibilità elettorale è dovuta al prevalere della politica digitale su quella reale. Una comunicazione iper-semplificata, sensazionalistica, ammiccante, ricalcata su quella pubblicitaria e soprattutto rivolta ad un pubblico fedele che vuole leggere quello che sa già, e cioè che: i politici sono tutti corrotti e malvagi e che Grillo ha le soluzioni per tutto, e che il Movimento 5 Stelle amministra in maniera egregia le città in cui è al governo. La propaganda mediale e in particolare digitale del Movimento 5 Stelle è capace di produrre una dimensione immaginaria del proprio ruolo nella scena politica. Nella realtà, gli obiettivi politici del Movimento 5 Stelle non sono fatti per essere realizzati; sono polemici, senza un programma politico concreto e con il solo scopo di suscitare l'avversione per gli altri partiti (che non si preoccuperebbero dei problemi della gente). Non c'è l'obiettivo di modificare, attraverso un pensiero politico consolidato, la situazione sociale ed economica. Sono proposte politiche che potrebbero avere un seguito, ma nelle quali emerge un profondo dilettantismo e, peggio ancora, l'assoluta indifferenza di portarle avanti. Questa legge elettorale è contro il Movimento 5 Stelle e a tutti gli altri va bene? Ma non diciamo sciocchezze! Contro il Movimento 5 Stelle c'è solo il fatto che, rifiutando *a priori* ogni compromesso tattico con le altre forze politiche, nessuna delle loro proposte ha la possibilità di essere realizzata, a meno di non riuscire ad avere la maggioranza assoluta nei due rami del Parlamento alle prossime elezioni e, non avendo più visto sollevare in Aula fogli con scritto "51 per cento", credo che non ci credano neppure i più ottimisti o fanatici Andremo quindi a votare con questa legge elettorale e l'estraneità del Movimento 5 Stelle alla politica gli permetterà di alimentare l'aura di partito dei veri cittadini e degli onesti, evitando le prove imposte dal mondo reale, o minimizzandole con la propaganda quando si rivelano fallimentari. La questione seria è che l'ascesa di Grillo ha coinciso con la sparizione di qualsiasi opzione di sinistra dalla scena politica italiana. Il Movimento 5 Stelle è il sintomo, non la causa. I Cinquestelle hanno attirato gli elettori che non sopportavano più il narcisismo salottiero dei *leader*, i loro *slogan* vuoti e ciò che a suo tempo ha deluso anche me, cioè la mancanza di proposte sul lavoro, la giustizia, l'ambiente, la scuola e quant'altro. La politica si affidava ai magistrati e molti di noi si sono rivolti verso Grillo. Qualsiasi sia la legge elettorale (e - ripeto - questa è favorevole al Movimento 5 Stelle, se non altro perché hanno un tema forte per fare campagna elettorale, parlandone male e portando gente davanti al Senato a manifestare contro) una cosa con cui dovremo comunque fare i conti è la tentazione di affidare il comando a uomini soli, in diretta comunicazione con i loro popoli, che è rispuntata in Occidente. Questo è il vero pericolo che dovremo spiegare perché sul disinteresse della democrazia politica nascono i populismi autoritari del nostro tempo. Signora Presidente, devo confessare una difficoltà. Ho tentato di preparare un intervento strutturato, ma mi sono trovato ad incontrare un limite mio. Io non riesco a ragionare su qualcosa di irragionevole. Farò allora alcune considerazioni Per l'insieme della valutazione su questo disegno di legge, mi riconosco nell'intervento di ieri del collega Tocci, negli inutili emendamenti e nell'inutile lavoro

estero. Negli anni passati il tema di discussione sulla modifica, da fare o non fare, alla Costituzione al fine di prevedere il collegio estero era stato proprio questo. Il compromesso che tutte le forze politiche costruirono all'epoca prevedeva un numero chiuso di parlamentari e che questi parlamentari dovessero risiedere nel collegio estero. Era il riconoscimento di una rappresentanza di comunità che vivono una realtà diversa da quella nazionale, con l'altra giusta correzione che questi eletti non devono avere lo stesso peso che hanno i cittadini che risiedono permanentemente in Italia. In effetti, se noi facessimo il rapporto numerico,

Nessun italiano all'estero nutre, neanche nell'anticamera del cervello, una idea del genere. Noi pensavamo, infatti, che il nostro ruolo qui dovesse essere un altro: quello di rappresentare una comunità e non solamente delle parti politiche.

si badi bene, evitando il rischio di candidature ad effetto che rischierebbero di svuotare la ragione stessa dell'istituzione della circoscrizione estero, portando all'elezione di personalità, magari rinomate, ma con nessun legame rispetto ai propri rappresentanti e difficilmente in grado di garantire quello specifico tipo di rapporto rappresentativo che la modificazione costituzionale, piaccia piaccia o non piaccia, ha inteso rendere possibile per dare voce alle specialissime istanze dei cittadini residenti lontano dall'Italia e per favorire il mantenimento di legami che la distanza rende più difficile da coltivare: fini per i quali sono, appunto, utili e giustificati garanzie e requisiti particolari nel pieno rispetto della Costituzione e di una interpretazione vuoi letterale vuoi sistematica, degli articoli 3, 48, 51, 56 e 57 della Costituzione». Questo era lo spirito. E con questo spirito gli italiani all'estero hanno accolto il collegio estero cercando di dare un loro contributo. Oggi tutto questo viene distrutto - non modificato

Rita Pavone, che è residente in Ticino. Dopo le elezioni, siamo andati a contare i voti e ha avuto venti volte meno le mie preferenze. Abbiamo avuto anche l'onore di avere come candidato un principe, quello che ha

Verdini". Il nome di Verdini non è uscito adesso; negli ambienti degli italiani all'estero, dopo il primo abbraccio di Verdini a Renzi, Renzi, incominciò a circolare questa voce. Io l'ho presa per "intossicazione" e non come informazione perché non ho mai dato seguito a quelle voci, però adesso incominciano ad arrivare altre informazioni, e questo potrebbe essere uno dei motivi. Dubito che il senatore Verdini abbia bisogno di candidare se stesso

Ci sforziamo altresì a far mantenere questo legame ai nostri figli, ai nostri nipoti perché abbiamo il difetto di essere affettivamente legati all'Italia. all'Italia. La presenza di parlamentari esteri nel Parlamento italiano - l'ho detto più volte e lo voglio ripetere qui - non è un interesse primario della nostra gente: dovrebbe essere, e secondo me è, interesse dell'Italia.

cinque fiducie, un voto finale, i tempi ristretti, gli emendamenti scritti e da buttare, credo che un po' di indulgenza, plenaria o parziale, da parte della Presidenza potrebbe esserci.

Credo che anche mio padre, che andò in Svizzera a scaricare il carbone, avesse un cervello. Tutti gli italiani all'estero hanno un cervello è servito all'Italia: pensiamo agli operai della Volkswagen e delle miniere belghe che hanno rimandato soldi in Italia per decenni per permettere anche il miracolo economico e costruire e sviluppare le zona depresse di questo Paese. Quei cervelli servono oggi quando sono ricercatori e quando sono capitani d'industria

Questa modifica costituzionale, Presidente, è stata copiata da altri Paesi; è l'unica cosa che la Francia ha copiato all'Italia. Immaginate: la Francia che copia qualcosa all'Italia; eppure lo ha fatto. Altri Paesi la stanno valutando e noi l'abbiamo distrutta. L'abbiamo distrutta, in parte per responsabilità nostra, dei residenti all'estero, ma anche perché i partiti hanno sempre e solo visto nei collegi esteri una "riserva indiana" di 18 seggi, da prendere in qualsiasi condizione e a qualsiasi costo. Questo è inaccettabile.

la governabilità è garantita dalla politica: in in Francia hanno eletto un Presidente della Repubblica e quando questo si è trovato a governare con un Parlamento di un altro colore, è stata garantita la governabilità del Paese. È la politica, non la legge elettorale, che garantisce la governabilità. Se non siamo stati in grado di garantire la governabilità di questo Paese è responsabilità della politica e sicuramente non della legge elettorale.

«Se vi è piaciuto Chernobyl, non perdetevi Creys-Malville», che era una centrale nucleare vicino a Ginevra. Con il clima che stiamo ricostruendo, mi piacerebbe scrivere su una maglietta: «Se vi è piaciuto il 4 dicembre, non perdetevi le prossime politiche».

è chiaro che il vostro intento è quello di salvaguardare il sistema di potere. Un sistema di potere che non può subire alcuna microsbavatura. Avete scelto di violentare per l'ennesima volta i cittadini italiani tramite la creazione di una legge elettorale anticostituzionale, imponendo il silenzio e denigrando

Non si può imporre una legge elettorale con il voto di fiducia ad un Governo non eletto, creato e messo in piedi per scelte di potere e casta. Avete il terrore dei cittadini. Avete il terrore che i cittadini sovrani possano scegliere i propri rappresentanti in Parlamento. Avete perso il lume della ragione scrivendo un testo di legge che ha in sé numerose incongruenze. Pensate che una legge elettorale che scippi il voto ai cittadini possa assicurarvi ancora una lunga vita di potere? Siete convinti che i cittadini siano il male peggiore di questa Nazione, offesa e vituperata nel territorio, nelle coste, nei fiumi e nei mari? Ebbene, vi sbagliate. I cittadini sanno e sapranno scegliere.

il collega Collina che ieri ha affermato che la legge elettorale ha l'obiettivo di trasferire in seggi il voto di 47 milioni di italiani e, come secondo obiettivo, garantire governabilità e rappresentatività. Questa legge non lo fa, senatore Collina, le do questa notizia.

Semplicemente perché il Movimento 5 Stelle e Forza Italia hanno chiesto che la legge elettorale fosse uguale in tutta Italia.

parla a vanvera, esclusivamente per arraffare, come ha fatto in questi anni, in tutte le maggioranze cui ha partecipato. Egli non risponde alla Nazione, ma risponde esclusivamente a se stesso e basta. *(Applausi

mettere in sicurezza il sistema e le istituzioni.

PD e Forza Italia - e alle varie *lobby*. Siamo contro questo sistema e siamo invece a favore delle istituzioni. Sì, noi ci crediamo nelle istituzioni, tanto che ci siamo spesi in occasione della riforma istituzionale per salvare il Senato.

Non accetto assolutamente lezioni da chi si professa "professorone" e ritiene di aver fatto parte di un partito che non lo rappresentava. Ritengo che ad una persona che ha ragion d'essere in quanto "ex" e non in quanto persona non si debba dare nemmeno una singola risposta.

Siamo ancora qui a dirvi le stesse parole che abbiamo già usato altre volte, perché state nuovamente e sfacciatamente profanando le istituzioni democratiche di questo Paese. Non è bastato un *referendum* bocciato dal 60 per cento degli italiani, perché oggi siamo in Aula per discutere la terza legge elettorale di questa legislatura. Voi del Partito Democratico, il vostro Governo e tutti quelli che lo sostengono sapete fare soltanto due tipi di leggi: quelle incostituzionali e quelle che servono a voi stessi. *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Purtroppo per gli italiani, questa legge truffa, il Rosatellum, fa entrambe le cose. Seconda fiducia. Vergogna perché siete ubriachi di Rosatellum, una legge elettorale annacquata che noi non vogliamo bere! Siamo ancora qui a dirvi le stesse parole che abbiamo già usato altre volte perché state nuovamente e sfacciatamente profanando le istituzioni democratiche di questo Paese. Non è bastato un *referendum* bocciato dal 60 per cento degli italiani perché oggi siamo in Assemblea per discutere la terza legge elettorale di questa legislatura. Voi del Governo, del Partito Democratico e tutti quelli che lo sostengono sapete fare solo due tipi di leggi: quelle incostituzionali e quelle che servono a voi stessi e, purtroppo per gli italiani, questa legge truffa, il Rosatellum, fa entrambe le cose. *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Terza fiducia. Vergogna perché siete ubriachi di Rosatellum, una legge elettorale annacquata che noi del Movimento 5 Stelle e i cittadini non vogliamo bere! Siamo ancora qui a dirvi le stesse parole che abbiamo usato altre volte perché state nuovamente e sfacciatamente profanando le istituzioni democratiche di questo Paese. Non vi è bastato un *referendum* bocciato dal 60 per cento degli italiani, perché oggi siamo in Assemblea a discutere la terza legge elettorale di questa legislatura. Voi del Partito Democratico, il vostro Governo e tutti quelli che lo sostengono sapete fare solo due tipi di leggi: quelle incostituzionali e quelle che servono a voi stessi e, purtroppo per gli italiani, questa legge fa entrambe le cose. Quarta fiducia. Vergogna perché siete ubriachi di Rosatellum, una legge elettorale che noi non vogliamo bere! Siamo ancora qui a dirvi le stesse parole che abbiamo già usato altre volte perché state nuovamente e sfacciatamente

Voi del Partito Democratico sapete fare solo due tipi di leggi: quelle incostituzionali e quelle che servono a voi stessi e il Rosatellum fa entrambe le cose!

Siamo ancora qui a dirvi le stesse parole che abbiamo già usato molte altre volte perché state nuovamente e sfacciatamente profanando le istituzioni democratiche di questo Paese.

voi del Partito Democratico siete in grado di fare soltanto due tipi di leggi: quelle incostituzionali e quelle che servono a voi stessi e il Rosatellum, questa legge elettorale truffa, purtroppo per gli italiani, fa entrambe le cose! Vergogna!

perché forse vi siete accorti che, parlando, qualcuno vi può ascoltare e fare le proprie considerazioni ed essere informato». Si sa che l'informazione in questo periodo, periodo, per la maggioranza e per questo Governo, non è una cosa da tenere in considerazione, perché può diventare pericolosa. Presidente, a questo punto farei un richiamo al Regolamento - lo dico seriamente

negli ultimi anni sono state proposte leggi come il Porcellum (incostituzionale); la riforma Fornero (un disastro);

Parliamo ancora di sblocca Italia, quindi praticamente di trivelle selvagge: basta venire in Basilicata per capire cosa è successo anche su questo fronte. In tutto questo panorama, come se nulla fosse successo negli ultimi

Peccato che dopo poche settimane, una volta scongiurato il*referendum*, hanno riproposto - forse in forma ancora peggiore - i *voucher*.

senatori di parlare sulla legge elettorale, questo dovrebbe essere un problema per tutti i senatori, perché questa si chiama democrazia. Se non si risponde, praticamente mai, alle interrogazioni parlamentari, parlamentari, questo è un problema di tutto il Senato, di tutti i senatori e di tutti i parlamentari. Guardate che questo è lo specchio del Paese.

sostanzialmente è già stato deciso tutto; Matteo Renzi, Silvio Berlusconi e Verdini hanno deciso come cercare di proteggersi e poter tornare qui. Noi continuiamo

secondo il Partito Democratico? Il dibattito sterile, del tipo: «Sì, lasciateli parlare, lasciateli dire, tanto poi facciamo noi». È la stessa cosa che è stata fatta con la riforma costituzionale. Poi, fuori di qui, c'è stata la sentenza da parte dei cittadini, che li ha voluti perdenti. Ora, contrariamente ai miei colleghi, intervengo per dire che non dire che non mi sento affatto scoraggiata, perché confido nei cittadini, in quei cittadini che ricorderanno. Ricorderanno che il Partito Democratico ha regalato diversi miliardi di euro alle banche, senza provvedere ai beni degli ultimi.

Ricorderanno la buona scuola, con gli insegnanti "deportati" e una didattica vecchia;

altro che Rosatellum: sono certa che vi daranno una bella batosta e finalmente saranno loro a mandarvi a casa. Per noi ha poca importanza chi tornerà qui, se sarà Barbara Lezzi, se sarà Sara Paglini, se sarà Manuela Serra o Vincenzo Santangelo: l'importante è che torni qui sempre più numeroso il Movimento 5 Stelle. Una cosa è sicura: andando a votare le accozzaglie che si andranno a formare, il cittadino non saprà chi manderà qui a rappresentarlo; con questa serie di slittamenti andranno un po' giù e un po' su, la maggioranza deciderà per tutti e non si saprà con precisione quale sarà la lista che prenderà più voti e che avrà più rappresentanti. Persino la Lega dovrà cedere qualche voto del Veneto magari alla Sicilia, perché è stato creato qualcosa di veramente diabolico. Quello che è certo

grande, potente voto utile che si potrà dare con questa orribile legge elettorale, che poi in seguito verrà nuovamente bocciata. Ma voi siete abituati ai fallimenti. Il Partito Democratico insieme a Forza Italia negli ultimi vent'anni non ha fatto altro che aumentare sempre le tasse, anche

lo sanno ed è questo che mi interessa. Avete solo qualche altro mese per fare regalini alle banche, a qualche *lobby*, per cercare di giustificarvi per quello che combinate. Per il resto, sarà un futuro del Movimento 5 Stelle, in cui il cittadino sarà finalmente padrone a casa sua e sarà ripristinata la democrazia.

mi sono chiesto fino a qualche minuto fa se fare o no questo intervento, perché la sua efficacia all'interno del Parlamento è pressoché nulla, ormai lo abbiamo capito: in questo Parlamento non si può discutere, non si può entrare nel merito delle questioni. In Commissione siamo stati bloccati, siamo stati impossibilitati ad apporre eventuali modifiche. In Aula i tempi sono stati contingentati,

Quella che si sta facendo oggi è una farsa, perché è una discussione su una fiducia; anzi no, signor Presidente, su una fiducia quintupla,

il testo che è stato votato alla Camera non è lo stesso che sarà votato qui in Senato. Questo è un dato di fatto oggettivo. Questo sistema non consente di modificare un errore fatto alla Camera, perché il Senato per questioni regolamentari non può intervenire su quello che è stato fatto alla Camera. A quel punto che cosa fai? Pensi che gli arbitri istituzionali, quelle figure che dovrebbero essere sopra le parti,

legge che non concede all'elettore la possibilità di scrivere un nome e di scegliere il proprio rappresentante, una legge dove il voto dell'elettore viene trasportato magicamente da una Regione all'altra, per andare a saziare chissà quale alleanza elettorale fatta in un'altra Regione, non è una legge democratica

Un Parlamento che partorisce una, due o tre leggi incostituzionali non è un Parlamento degno di questo nome. I senatori e i deputati che fanno parte di questo Parlamento non sono degni di essere chiamati onorevoli.

cravatta)*. Però se c'è una legge incostituzionale - e tutti sappiamo che è incostituzionale - non c'è un modo democratico di poterne discutere! Questo posto è il contrario di tutto. Abbiamo cercato di porre la questione alla vostra attenzione e ieri mi sono anche aggrappato a uno dei banchi del Governo. Mi hanno messo le mani addosso, perché questa cosa non si può fare.

allora fatto con tutta la forza che avevo e continuerò a farlo fino all'ultimo istante in cui sarò dentro le istituzioni, ma anche fuori dalle istituzioni, perché il *modus operandi* di questo Parlamento non è sano. Non è sano per voi, ma soprattutto per gli italiani. *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Non indietreggiate di un millimetro e vi aspettiamo questo pomeriggio fuori in piazza, perché stare qua dentro non serve assolutamente a nulla.

al di fuori da ogni correttezza istituzionale, che impedisce, di fatto, una discussione articolata, seria e approfondita da parte dell'Assemblea su una norma che sta alla base del funzionamento delle nostre istituzioni. Una violenza al Parlamento segno, al tempo stesso, di protervia e arroganza, ma anche di debolezza di chi incapace di svolgere una corretta discussione non può fare altro che usare le armi della prevaricazione. Appare anche evidente che la scelta di porre la questione di fiducia sia rivolta non solo verso i Gruppi parlamentari che stanno contrastando questa riforma elettorale profondamente sbagliata, ma ancor di più a silenziare le voci di dissenso presenti nella stessa maggioranza e, in modo particolare, nel Partito Democratico. Con questa scelta, inoltre, il Governo è venuto meno all'impegno assunto dal Presidente del Consiglio all'atto del suo insediamento e cioè di non interferire nella discussione parlamentare sulla nuova legge elettorale. Il presidente Gentiloni Silveri è il primo Presidente del Consiglio a porre la fiducia su questo tema in entrambe le Camere; un triste primato e una invasione di campo del Governo in una materia parlamentare che non sarebbe concepibile in alcuna grande democrazia, per di più a pochi mesi da nuove elezioni. È un atto, questo, estremamente grave e che potrà avere forti ripercussioni nei rapporti tra le forze politiche, nonché sull'*iter* dei futuri provvedimenti. In realtà, questa riforma non ha l'obiettivo di dare al Paese un'adeguata legge elettorale che garantisca una maggioranza di Governo, favorisca le aggregazioni e riconsegni ai cittadini la scelta dei parlamentari. L'obiettivo, invece, è difendere alcune forze politiche, in particolare il Partito Democratico e Forza Italia, e salvaguardarne la presenza parlamentare, in una sorta di arrocco del sistema che segnerebbe, un'altra volta, la distanza dal Paese reale, dalle sue ansie e preoccupazioni. un'operazione tutta politica di difesa dell'esistente. Con il provvedimento in discussione nasce perciò nelle Aule parlamentari, dopo essere nato nei retrobottega della politica, il Governo Renzi, Verdini, Berlusconi. Questa legge elettorale è fatta proprio per cercare di garantire questa indigeribile ammucchiata nella prossima legislatura. Scendendo nel dettaglio della riforma, come hanno già fatto diversi colleghi del mio Gruppo, essa mostra limiti e incongruenze che ne fanno una pessima legge elettorale, incapace di rispondere alle necessità di rappresentatività e governabilità che da tempo sono diventate più che mai indispensabili per il funzionamento del nostro sistema politico e istituzionale. Per quanto riguarda la parte maggioritaria, che eleggerà un terzo dei futuri parlamentari, essa consente il formarsi di apparentamenti estemporanei e raffazzonati nei diversi collegi: invece di avere una coerente coalizione di forze politiche, legate da un comune programma elettorale, un unico simbolo, ci troveremo di fronte alle alleanze più varie, spesso contraddittorie e legate soltanto dagli interessi di piccoli e grandi sistemi di notabili locali. una vera regressione istituzionale e politica, buona per rappresentare appunto i potentati locali e non certo per saldare quel necessario rapporto tra eletto, territorio e cittadini. Come è noto, il maggior numero degli eletti arriverà dalla parte proporzionale. Essi, tuttavia, verranno determinati nei fatti dal voto maggioritario con un discutibile meccanismo. A ben guardare, l'elettore non sarà libero di scegliere il voto nella parte proporzionale: non esiste la possibilità di scegliere un candidato nella parte maggioritaria e una lista in quella proporzionale che non siano apparentati, come accade nel sistema elettorale tedesco, spesso citato a sproposito - insisto sul punto - da chi difende questo sistema. In questo modo, quindi, si limita la possibilità di scelta dell'elettore, costringendolo nei fatti a un'opzione unica sia per la parte maggioritaria che per quella proporzionale. Con il ricorso alle liste bloccate, poi, si impedisce ancora una volta ai cittadini di scegliere il parlamentare. A ciò si accompagna il possibile ricorso alle candidature multiple che, in un sistema politico fatto sempre più da forze sottoposte a un sistema afflitto da leaderismo, si traduce nel fatto che i vertici dei partiti avranno l'assoluto controllo su coloro che saranno eletti, determinandoli prima ancora che si vada alle urne. Tutto ciò segnerà un ulteriore distacco - mi rivolgo soprattutto ai colleghi del Partito Democratico su questo punto - tra il Paese e il sistema politico, aggravando la già pesante e profonda sfiducia nelle istituzioni, presente in larga parte dell'opinione pubblica. Sempre sulla parte proporzionale, merita attenzione il furbesco trucco inventato con il sistema degli sbarramenti elettorali. Lo sbarramento al 3 per cento si accompagna all'introduzione di un'ulteriore soglia dell'uno Infatti, si prevede che le liste che non raggiungano il 3 per cento, ma con un risultato superiore all'uno, concorrano in ogni caso alla determinazione della cifra elettorale delle forze apparentate. punti il nostro Gruppo Articolo 1 - Movimento democratico e progressista ha presentato pregiudiziali di costituzionalità e certamente la Corte costituzionale avrà modo di valutare la coerenza della normativa con il nostro ordinamento costituzionale. In ogni caso, si tratta di una furbata che tra l'altro vanifica l'introduzione della soglia di sbarramento come deterrente alla frammentazione della rappresentanza parlamentare. Un ultimo aspetto, signor Presidente, merita la nostra attenzione: l'introduzione nella legge dell'indicazione del *leader* della lista. A parte il fatto che essa protrae l'equivoco presso l'opinione pubblica che si vada, in qualche modo, all'elezione diretta del *Premier*, cosa del tutto al di fuori del nostro dettato costituzionale, ci si ritrova in questo caso, come già segnalato da altri colleghi, nella grottesca situazione in cui un cittadino voterebbe per una coalizione formata da *leader* diversi e con diversi programmi elettorali. Signor Presidente, è del tutto evidente quindi che questa legge ha in sé diversi e contradditori aspetti, che non ne fanno in alcun modo quella legge elettorale necessaria per il buon funzionamento del nostro sistema. Essa invece, come detto, rappresenta lo stanco espediente di alcune forze politiche per mantenere le proprie posizioni e per chiudersi rispetto alle esigenze della società italiana. Una legge, inoltre, che chiude la porta alla prospettiva di avere coerenti e solide coalizioni elettorali e che rappresenta, da parte del Partito Democratico e del suo capo, una scelta di campo netta: rompere con la sinistra e il suo elettorato. In questo modo si rinuncia alla prospettiva di ricostruzione di un centrosinistra che abbia a cuore le sorti della nostra democrazia e i bisogni dei cittadini. Chi oggi, con testarda ottusità, ha percorso la strada di una scelta sbagliata e nociva avrà la responsabilità di una rottura tra le forze di progresso alle prossime tornate elettorali, sia in quella nazionale, come probabilmente in quelle che si svolgeranno in diverse Regioni. Si tratta, per concludere, di una scelta di autodifesa di un pezzo del sistema politico, priva del respiro e della lungimiranza necessaria in questa fase storica. Un espediente che si propone di chiudere a riccio il sistema politico-istituzionale esistente, cercando al contempo di eliminare tutte le voci dissenzienti e che ha come unico obiettivo saldare e garantire il patto consociativo tra il Partito Democratico, a guida renziana, e Forza Italia, tra Renzi e Berlusconi, con la copertura logistica di Verdini, costruito in questa legislatura e che si vuole protrarre nella prossima.

*(PD)*. Signor Presidente, colleghe e colleghi, vorrei aggiungere alcune considerazioni a quelle che gli altri colleghi eletti nella circoscrizione estero hanno illustrato nei loro interventi. interventi. Se consideriamo questo disegno di legge al di là delle logiche di partito, secondo me esso costituisce un passo nella direzione giusta. Sono un convinto sostenitore dell'importanza della rappresentanza parlamentare territoriale e la legge elettorale che ci accingiamo a votare introduce collegi uninominali e listini brevi. Non possiamo negare che ciò costituisca un passo in avanti rispetto al passato. Penso però che sarebbe stato bene andare oltre, prevedendo anche l'obbligo della residenza dei candidati nelle circoscrizioni in cui si presentano. I cittadini avrebbero avuto la garanzia di eleggere persone che vivono nelle loro comunità, che conoscono il territorio e che possono quindi essere i migliori interpreti delle loro esigenze. Purtroppo, pochi degli interventi che mi hanno preceduto hanno toccato questo aspetto della legge. Noto invece delle contraddizioni all'interno della legge. Una di queste è il fatto che la circoscrizione estero era l'unica realtà di rappresentanza diretta di candidati collegati al territorio. Purtroppo, a causa di quanto previsto dall'articolo 6, non lo sarà più. Non mi convince la giustificazione della norma che permette ai residenti in Italia di candidarsi nella circoscrizione estero. Oserei dire che non esiste alcuna giustificazione logica. Da un lato un passo in avanti, con i collegi uninominali in Italia, e dall'altro due indietro, permettendo a chi risiede in Italia di candidarsi a rappresentare gli italiani nel mondo. Mi sembra una grande contraddizione. Vi è un'altra contraddizione, signor Presidente, sempre nell'articolo 6 ove è previsto che non sono candidabili i cittadini italiani che negli ultimi cinque anni hanno ricoperto cariche elettive in uno Stato estero, che per gli iscritti all'AIRE e il loro Paese di residenza. Anche in questo caso non riesco a capirne la logica. Qual è la differenza fra un cittadino italiano che viene eletto in un consiglio comunale in Italia ed un cittadino italiano che viene eletto in un consiglio comunale all'estero? Se crediamo nei valori della politica, in entrambi i casi si tratta di cittadini italiani che hanno messo a disposizione il loro tempo, il loro impegno, le loro persone, per le comunità in cui vivono. Non capisco come possano essere trattati in maniera diversa a seconda del luogo in cui vivono. Questa sarà un'altra contraddizione che verrà introdotta dalla nuova legge. Avevamo presentato un emendamento per eliminare queste contraddizioni. Purtroppo il ricorso al voto di fiducia ci impedisce di approfondirne le ragioni e di invitare l'Assemblea a considerarle. Io credo nell'attuale Governo, l'ho sempre sostenuto e continuerò a sostenerlo, anche con i voti di fiducia di oggi che daranno all'Italia una nuova legge elettorale, necessaria per il Paese.

anzi, mi lasci dire che abbiamo perso un'ottima occasione per discutere seriamente della rappresentanza parlamentare degli italiani nel mondo e del loro contributo per lo sviluppo ed il futuro del nostro Paese. In conclusione, signor Presidente, avremo una nuova legge elettorale che, malgrado non sia la soluzione ottimale, introduce regole uniformi per Camera e Senato, collegi uninominali e listini ridotti, ma toglie anche l'unica vera rappresentanza parlamentare territoriale, permettendo ai residenti in Italia di candidarsi all'estero e contraddice lo spirito della riforma costituzionale che ha permesso la rappresentanza in parlamento agli oltre 4.000.000 di italiani nel mondo. Mi creda, come affermava prima il senatore Micheloni, a perdere non saranno coloro che vivono all'estero ma sarà l'Italia che forse, anche per colpa nostra,

Signor Presidente, noi del Movimento 5 Stelle, in questi anni, ci siamo sentiti accusare di essere antipolitica ed antisistema, accuse che rigettiamo al mittente. La vera antipolitica e il vero antisistema democratico siete voi, voi della maggioranza e mi spiace spiace per il presidente Grasso, ma anche lui si è reso complice di questo antisistema democratico. Dopo il *referendum* del quattro dicembre il popolo italiano si aspettava una presa di coscienza da quei parlamentari che avevano votato una riforma della Costituzione bocciata dai cittadini. Invece nulla. Come vi dissi un giorno: avete abbassato il capo al capo. Siete abituati a scegliere, se vi conviene, il meno peggio. Mi auguro non lo abbiate fatto anche quando vi siete sposati. Noi vogliamo il meglio per questo Paese, vogliamo dei parlamentari onesti e liberi. State mentendo ai cittadini. Il PD si presenterà in coalizione con i vari Idv, Mastella e altri per raccattare qualche voto in più, per poi confluire nella coalizione preferita: PD-Forza Italia con contorno di Verdini e Salvini. Come fate a non vergognarvi? Io credevo che in quest'Assemblea - di alcuni avevo anche stima - ci fossero persone sane, e e invece mi devo ricredere. In questi giorni sono stata in Sicilia, ho parlato con i siciliani e mi sono resa conto che i mafiosi non sono in Sicilia ma qui e il cinque novembre noi abbiamo la possibilità di dare un segno al Paese, partendo dalla Sicilia, Sicilia, per esprimere un voto consapevole e mandare a casa quella coalizione di partiti, quell'accozzaglia di parlamentari, che attualmente si stanno mangiando il Paese e questa legge nazionale non fa altro che riconfermare quell'accozzaglia di parlamentari che veramente dovrebbero andare a casa.

mi rivolgo ai pochi, pochissimi, rimasti in quest'Aula per questo "Zittamento", anziché Parlamento, per citare il collega. Mi rivolgo, in particolare, a chi ci ascolta da casa per ricordare alcuni punti. Chi ha urlato nelle piazze che il Porcellum era una schifezza incostituzionale? Noi, il Movimento 5 Stelle, da quel famoso V-*day*. Gli ignoranti costituzionali, i barbari costituzionali, gli incompetenti. Ma la Corte costituzionale Chi vi ha detto che la riforma costituzionale non avrebbe avuto il consenso del popolo? Noi, sempre gli incompetenti. E chi vi ha detto che l'Italicum era incostituzionale? Ve lo ricordate o lo avete rimosso? Sempre noi, quelli cui date degli incompetenti. Ve l'avevamo detto che l'Italicum era incostituzionale. Chi vi ha detto che dovevate fare una legge elettorale anche per il Senato? Vogliamo ricordare chi è responsabile di avere fatto una legge elettorale solo per una Camera? Ve lo dicevamo allora.

Chi vi sta dicendo oggi che state facendo una legge elettorale truffa, una legge elettorale incostituzionale? Sempre noi, sempre gli incompetenti, che continuano a ripetere le stesse cose e alla fine hanno ragione. Invece, i professoroni al libro paga del Partito Democratico

Due leggi elettorali sbagliate. Ma non c'è due senza tre e voi, imperterriti, proseguite a fare la terza legge elettorale da buttare nel cesso! *(Applausi ai recidivi non si dà la condizionale, non si dà la pena sospesa. I recidivi si sbattono direttamente in galera. Voi, invece, state ripetendo lo stesso errore: siete colpevoli di truffa aggravata nei confronti dei cittadini, aggravata dalla recidiva!

Ripeto che siete colpevoli di reato di truffa aggravata dalla recidiva nei confronti dei cittadini italiani. Ma gli italiani sono più intelligenti e non ci cascheranno, anche perché ci sarà qualcuno che denuncerà tutto questo. Così come abbiamo fatto in Sicilia, con Giancarlo Cancelleri, che ha pubblicato l'elenco degli impresentabili in entrambe le liste, del centrodestra

informazioni diffuse in queste ore è chiaro che Renzi sta liquidando il Partito Democratico; lo sta smembrando, come fa il liquidatore di un'azienda, per consegnarlo ai suoi acquirenti futuri, i cinesi di Forza Italia. Questo è ciò che sta facendo e voi lo state aiutando. Pensateci bene quando il Partito Democratico sarà tutto nelle mani di Berlusconi e Verdini!

qualche esempio. In una Repubblica parlamentare il prodotto legislativo dovrebbe uscire dall'unione della volontà delle persone che sono qua dentro. Non è così. Prevale sempre la maggioranza, e prevale al punto tale che la Presidenza dà costantemente ragione alla maggioranza, quindi nel 100 per cento dei casi, qualunque sia la materia del contendere. È statisticamente e probabilisticamente impossibile impossibile che ciò avvenga, ma è così. Perché questo? Perché la Presidenza si gira a sinistra, nella buca del suggeritore, e dalla buca del suggeritore gli arriva sempre l'indicazione giusta per dire che quanto sostenuto dall'opposizione è sbagliato, anche quando è controfattuale, come è successo ieri. Nel qual caso, vedo la Presidenza che, come un bambino capriccioso, dice no perché ormai ha deciso così e così si fa. Questa La parola democrazia in questo momento è diventata un insulto qua dentro, come la questione di fiducia che ancora una volta è stata posta. Del tutto legittima: la legge n. 400 del 1988 disciplina il modo in cui la potete porre, e di fatto la ponete. La procedura seguita è quella normale? Sì, avete anche rispettato l'articolo 72

la legge elettorale che sta al legislatore ordinario doveva essere figlia del tempo, e cioè, se mutano le esigenze all'interno di una Nazione le leggi elettorali devono essere sufficientemente flessibili. Quindi, anche se un ordine del giorno dell'Assemblea costituente diceva che il sistema migliore era quello proporzionale (e lo credo bene che è

Per questo fu bocciato il premio di maggioranza. Comprimere la libertà dell'elettore vuole anche dire che il suo voto non va nel bersaglio che si vuole colpire. Dove sta il problema? Sta nel fatto che quando un elettore avrà le due schede elettorali e poi si troverà nell'urna anche il tubetto della vasellina - perché questo provvedimento ha il connubio non saprà più esattamente cosa sta votando; peggio ancora, si troverà a votare qualcosa a naso turato. Supponiamo che Forza Italia e la Lega decidano di fare questa accoppiata questa accoppiata e che un elettore della Lega non sopporti il candidato uninominale di Forza Italia perché, per esempio, la Lega vuole uscire dall'euro, mentre Forza Italia vuole fare il contrario. contrario. Nel momento in cui egli votasse e mettesse una x sulla Lega, il suo voto andrebbe inevitabilmente a Forza Italia e quindi l'elettore non potrebbe scegliere liberamente. Di conseguenza, o rinuncia al suo diritto di votare, perché dice che queste condizioni non gli piacciono, oppure accetta qualcosa che non appartiene alla sua volontà. Questi sono forse il peggior trucco e la peggior truffa che voi potevate fare agli italiani; è la massima compressione del diritto di voto. Costringete qualcuno ad autolimitarsi o, addirittura, a rinunciare o a votare ciò che non gli piace, perché quello è il piatto che gli avete preparato. Ritengo che su questo punto la Corte costituzionale si esprimerà.

È iscritto a parlare il senatore Chiti. Ne ha facoltà.

si apprestano a votare questa legge un po' *obtorto collo*, non certo perché persuaso che sia la giusta medicina per il nostro Paese, lacerato da interessi di parte e zavorrato dal debito pubblico, che ne è la conseguenza, ma perché consapevole che l'alternativa, lasciare cioè il Consultellum, sarebbe assai peggio. scopo della legge sarebbe quello di rendere omogenei i sistemi e i risultati elettorali tra Camera e Senato. In teoria questo dovrebbe aiutare la governabilità, non essendo più costretto l'Esecutivo a rincorrere due maggioranze diverse nelle due Camere.

Si tratta dunque di una chimera, ma l'aspetto ipocrita si manifesta nelle posizioni di coloro che oggi criticano il Rosatellum perché non garantirebbe la governabilità e, meno di un anno fa, contestavano la riforma costituzionale che, differendo le funzioni di Camera e Senato, invece la agevolava. La verità è che per una parte delle opposizioni, soprattutto per le sue numerose e super frammentate sinistre radicali, compito del Senato non dovrebbe essere quello di dare fiducia e contribuire al governo del Paese, ma quello di controllarlo, condizionarlo e, se necessario, ostacolarlo. Una visione legittima, per carità, ma che rivela una cultura politica che da tempo ha abdicato ad essere forza di trasformazione del Paese e si è rassegnata ad essere memoria nostalgica di una mancata rivoluzione in Italia, di cui abbiamo celebrato ieri il centenario con il bel discorso del senatore Tronti. Una cultura politica che nei suoi epigoni odierni appare oggi rancorosa e minoritaria, ossessionata, psicotica e autoipnotizzata dall'astio verso il Segretario del Partito democratico. Anche i membri del Movimento 5 Stelle sono altrettanto autoipnotizzati. C'è un ulteriore elemento di finzione e manipolazione della realtà che va denunciato, quello secondo il quale il Rosatellum sarebbe una legge volta ad introdurre un regime autoritario e antidemocratico; affermazione che, tra l'altro, fa a pugni con quella sulla governabilità che ho appena commentato. Certo, in questo dibattito ciascuno si sente ormai legittimato a dire tutto e il contrario di tutto. il Rosatellum introduce un sistema per due terzi proporzionale e per un terzo maggioritario. Il Mattarellum aveva proporzioni invertite e nessuno aveva mai eccepito: era per due terzi maggioritario e soltanto per un terzo proporzionale. Lo stesso dicasi per il cosiddetto Tedeschellum, la legge che fu in discussione a giugno, presso la Camera dei deputati, e che - a parole, ma non nel segreto del voto - anche il Movimento 5 Stelle aveva approvato. Ecco quindi l'ipocrisia di coloro che valutano di volta in volta la bontà di un sistema solo secondo le loro precise e personali convenienze elettorali. Ipocrita è anche la critica di chi lamenta la mancanza di un programma alla base della coalizione,

ma per una assai meno nobile discordia sulla candidatura a Capo dello Stato, concordata tra lo stesso Bersani e Berlusconi. Concludendo,

chi fa questa critica nulla obietta sul fatto che la legge attuale, se non venisse approvato l'Atto Senato 2941, di cui stiamo discutendo, sarebbe il cosiddetto Consultellum, una legge scritta con la tecnica delle sentenze additive. Quale sarebbe la maggiore legittimazione popolare della Corte costituzionale ad agire come legislatore, per di più in una materia che è sommamente politica come quella elettorale? Con il massimo rispetto per la Corte costituzionale, il nostro sistema delle fonti non la contempla tra i soggetti che hanno un potere di iniziativa legislativa e le sue sentenze sono state oggetto, da questo punto di vista, di molte critiche, anche a livello internazionale, per lo sconfinamento in un campo riservato al Parlamento. C'è molta ipocrisia in chi ha esultato per la fine dell'Italicum, che avrebbe assegnato agli elettori la scelta della maggioranza di Governo, che sarebbe risultata nota la sera stessa delle elezioni, e oggi si lamenta del fatto che tutti i Governi e le coalizioni saranno, con ogni probabilità, scelti dai partiti nell'ambito di trattative solo successive al voto. È ipocrita la critica di chi ritiene che non si dovrebbe intervenire in materia elettorale negli ultimi mesi della legislatura. Certo, questo è un principio condivisibile in astratto, ma è noto a tutti che non solo il Capo dello Stato, ma larghissima parte dell'opinione pubblica chiede a gran voce

voti segreti. Perché i cittadini, il popolo sovrano, non devono sapere come votano i rappresentanti su una legge massimamente politica come quella elettorale? Qui non c'è alcuna questione di coscienza, c'è soltanto da decidere che tipo di Paese vogliamo costruire per il futuro ed è giusto che ciascuno lo faccia a voce alta. Una volta il Movimento 5 Stelle e il suo guru, Beppe Grillo, avevano fatto della trasparenza la propria bandiera. Vediamo oggi che erano solo chiacchiere vuote, senza profondità di convinzione. Ben venga, dunque, il voto di fiducia, che porterà ciascuno di noi a doversi esprimere a voce e a testa alta con un sì o con un no, senza alibi, senza ipocrisie e neppure infingimenti.

La Commissione di Venezia, più volte citata, invita tutti gli Stati membri del Consiglio d'Europa a cambiare la legge elettorale almeno un anno prima delle elezioni stesse e in questo caso ciò non è avvenuto. Va detto però che una legge elettorale era stata approvata, ovvero l'Italicum, e abbiamo visto i risultati. Lo è nei modi

gli italiani ci hanno detto chiaramente che vogliono il bicameralismo paritario e quindi omogeneità tra le leggi elettorali della Camera dei deputati e del Senato. Poi c'è il fallimento, comunque,

Meno positivi sono i collegi plurinominali, perché non hanno preferenze, ma queste liste corte rendono riconoscibile agli elettori chi stanno votando

infine, un piccolo commento sulla questione della democrazia calpestata. Credo che la democrazia la stiamo vivendo in questo dibattito e la vedremo maggiormente quando i senatori presenti, rappresentanti dei cittadini, passeranno sotto il banco della Presidenza a dare il loro voto voto palese e libero - siamo senza vincolo di mandato - alla luce del sole. Tutti potranno giudicarci. Questa è la democrazia e la vedremo qua.

in questa Assemblea, nelle istituzioni. Io sono una cittadina normale e semplice che ha questa possibilità. Vorrei parlare a nome di chi è fuori, rifacendomi a una brevissima frase di Beccaria che scriveva: «Non vi è libertà ogni qualvolta le leggi permettono che, in alcuni eventi, l'uomo cessi di essere persona e diventi cosa». Parto da questo. Questa legge elettorale farà diventare le persone cose, perché se una persona non può esprimere il proprio voto liberamente e viene utilizzata per spostare la propria volontà, a secondo della convenienza del partito di maggioranza, non è più una persona libera: è una cosa. Per questo sono particolarmente orgogliosa di poter dire ciò in questa Assemblea. Vorrei ringraziare i cittadini che in questo momento sono nelle piazze e stanno facendo sentire la loro volontà di poter contare e di continuare a essere cittadini liberi in uno Stato democratico. Vorrei ringraziare i miei colleghi che da quattro anni e mezzo si stanno battendo in queste Assemblee

presenza importante e mi chiedo: lui, per tutti, cosa ne pensa di questa legge elettorale? Qual è l'urlo che gli viene dal cuore? davvero convinto che questa legge elettorale non sia una stortura della democrazia? Chiedo a voi un atto di coraggio, come lo sto facendo io in questo momento; l'atto di coraggio di poter dire veramente in libertà quello che pensate di quest'ennesima imposizione dall'alto di quattro persone che, fuori da queste Aule, hanno deciso anche per voi. Io potrò dire nella vita che ce l'ho messa tutta, in piena onestà, insieme ai miei compagni di lotta che sono qui e fuori da queste Aule. Non so se molti di voi potranno dire la stessa cosa né se potranno dire ai propri figli di aver consegnato un Paese libero nelle mani di chi verrà.

ringrazio tutti coloro che prenderanno atto di questo sopruso democratico, si presenteranno alle prossime elezioni e daranno il loro voto consapevole all'unica forza politica che continua con incessante energia

con questo intervento intendo motivare semplicemente le ragioni per le quali non voterò la legge elettorale in esame e, dunque, non parteciperò ai voti sulla fiducia né al voto finale sulla legge. È una distinzione dalle posizioni del mio Gruppo che mi pesa e pesa, ma che non posso evitare, perché aspetti rilevanti della normativa elettorale proposta sono in contrasto con le mie convinzioni; con quanto ho sostenuto dal 2005 in poi, quando venne approvato il cosiddetto Porcellum; con le battaglie che invano in questi anni con tanti altri ho portato avanti e anche per il fatto che sia stata posta la questione Di questa legge non mi convince la quota esigua dei colleghi uninominali. Impossibile andare oltre? Una prima e ampia intesa era stata raggiunta sul 50 per cento di collegi uninominali cento di proporzionale. Dunque, non era inverosimile quest'obiettivo. Ancora meno mi convince il voto unico, che impedisce una piena scelta da parte dei cittadini dei loro rappresentanti in Parlamento. Fu uno dei motivi che determinarono la mia decisione all'epoca di non votare neanche l'Italicum. Oggi questo *deficit*, che ha già prodotto una distanza enorme tra cittadini e istituzioni, mi appare non solo non risolto, ma in qualche modo aggravato. Non mi convince la pluralità delle soglie per l'accesso ai seggi, vizio tutto italiano: 3 per cento, 10 per cento per le coalizioni, ripescaggio dei voti di chi nelle coalizioni superi l'uno uno stimolo a moltiplicare le liste e a dar vita a schieramenti elettorali, non di Governo, come abbiamo già verificato. Non mi convince che si mantenga in vita l'ambiguità dell'indicazione del capo della forza politica, non è così e ha ragione il presidente Napolitano che, per primo, ha sollevato quest'aspetto. Non mi convince infine la previsione che si possa essere residenti in Italia e candidati nelle circoscrizioni estere: residenti a Fiesole, Castellammare di Stabia o ad Acireale e candidati in Canada, negli Stati Uniti o in Australia. Ho dubbi sulla correttezza costituzionale e certamente su quella della rappresentanza di un voto che, se dato solo al candidato in un collegio uninominale, verrà poi redistribuito anche alle liste che lo sostengono, in modo proporzionale ai consensi da esse ottenuti, al di là della volontà dei singoli cittadini. Si dice che

Questa funzione spetta certamente al Parlamento, ma non c'era e non c'è un'unica via d'uscita. Nella vita degli uomini e in quella politica gli stati di necessità si verificano a seguito di scelte, di impostazioni, quasi mai per caso. Per mesi si è perso tempo. Per mesi si è cullata proprio l'idea di andare a votare con le due leggi eterogenee, conseguenza delle decisioni della Consulta. Per mesi

non si potesse discutere nei Gruppi, nei partiti, come se fosse un fatto corporativo o settoriale. Penso che la fiducia posta dal Governo, alla Camera e al Senato, sia un serio errore. Mi colpisce la sottovalutazione della gravità di questa scelta, nascosta dietro la necessità di una legge. A questa richiesta, avanzata da taluni Gruppi della maggioranza - compreso il mio - e condivisa dall'opposizione di destra, sarebbe stato giusto rispondere con un no. Non era nel programma di Governo: lo aveva esplicitamente dichiarato alle Camere il Presidente del Consiglio nel suo discorso di insediamento. Non si giustifica per me la fiducia su leggi elettorali o sulla Costituzione. Sono principi astratti? No, sono valori da tenere fermi, oggi e domani, come è stato per ieri. In ogni caso, di questo errore ritengo quella del Governo la responsabilità minore. Più grande è quella dei Gruppi parlamentari che l'hanno voluta o condivisa, snaturando così lo stesso strumento della fiducia e dando un contributo al rafforzarsi di quella costituzione materiale che soffoca la Costituzione della nostra Repubblica. La fiducia che i Governi pongono, fin troppo spesso, per attuare il loro programma, e - va riconosciuto - anche per la mancata riforma delle nostre istituzioni, questa volta è stata invocata dal Parlamento per ridurre il suo ruolo, la sua funzione; limitare, anzi annullare il confronto al suo interno, addirittura su un tema fondamentale come la legge elettorale, giunta oltretutto alla sua approvazione al termine della legislatura. La fiducia si è così trasformata in una sorta di strumento per controllare voti segreti e ostruzionismo, una sorta di meccanismo alternativo e complementare a canguri, tagliole, eccetera. È difficile pensare che una maggioranza così ampia non sarebbe stata capace di sostenere o di orientare un confronto parlamentare serio e di battere eventuali sortite strumentali di quanti volessero assumersi la responsabilità di trucchi per imporre voti segreti non dovuti. Quello che ha più pesato - a mio giudizio - è piuttosto la volontà di far approvare a ogni costo questa legge elettorale prima del voto in Sicilia. Ancora una volta si è davanti a una sorta di ossessione per le scadenze, già vista in un recente passato, la cui rilevanza appare chiara soltanto nel ristretto ambito di una politica politicante, non per i cittadini. È difficile illudersi che i ripetuti voti di fiducia posti in questa legislatura dai Governi sulle leggi elettorali non costituiscano un grave precedente che peserà nel futuro della nostra democrazia. Il fine non giustifica i mezzi, non più almeno. Oggi una politica seria deve fondarsi su mezzi e fini, gli uni e gli altri validi. Nel dire questo non metto in sordina responsabilità che al Senato ha anche il Movimento 5 Stelle o, meno ancora, quelle di chi parla di "fascistellum": le parole hanno un significato preciso e violarlo è un inganno, non soltanto un abbaglio estremistico. Né posso condividere o non sottolineare le contraddizioni, le incoerenze di chi parla di trasparenza, di rifiuto del voto segreto e poi magari inventa possibili e strumentali voti segreti; sono accettabili scelte che bloccano, per interessi o propaganda di parte, il lavoro delle istituzioni alle quali si giura lealtà. Questo tipo di opposizione non è certo uguale al mio dissenso sulla legge elettorale: io non condivido obiettivi che perseguano il «tanto peggio, tanto meglio». L'Italia e le sue istituzioni non hanno bisogno di questi comportamenti. La mia collocazione non è quella di un non sostegno al Governo: sul suo programma, come sulla prossima legge di bilancio, il mio voto ci sarà. Oggi no, non può esserci, per i motivi che ho richiamato. Infine, faccio una considerazione conclusiva: non so se questa legge saprà dar vita a maggioranze di Governo stabili. Personalmente, ne dubito fortemente, ma non voglio fare qui previsioni sul futuro. Quello che vedo e che mi preoccupa, oltre alla questione irrisolta di una sovranità mortificata e di un Parlamento che non si confronta e non discute, è la divisione nel centrosinistra. Questa divisione, che mi auguro si possa superare, ma intanto si complica, lascerebbe ampi varchi a quel vento di destra che continua a soffiare forte in Europa. In Italia i rischi sono maggiori, non minori, perché c'è una destra partecipe del popolarismo europeo, ma che non è alternativa, bensì alleata di partiti lepenisti, ostili dunque all'Europa, all'euro, ai migranti. Voglio augurarmi che, nonostante questo passaggio non positivo, per la divaricazione che oggi si verifica anche sulla legge elettorale, restino aperte le porte per un dialogo sui programmi, per un'alleanza di centrosinistra da ricostruire prima che sia troppo tardi, prima cioè che la sua credibilità venga definitivamente meno e con essa venga meno la voglia di stare in campo, di partecipare, di impegnarsi di quei milioni di cittadini che ancora guardano a noi.

si parlerà di trasparenza dei partiti. E questo sarà un gravissimo e tragico errore di cui la maggioranza che approverà la legge sarà interamente responsabile. Partiamo dunque dalla Costituzione. l'articolo 49 «Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale». Secondo alcuni costituzionalisti, l'articolo 49 della Costituzione è quello che ha più bisogno di una legge di recepimento per esplicare i suoi benefici effetti. Per farlo, occorre però dare una corretta interpretazione alla clausola «con metodo democratico» contenuta nella sua formulazione. Il dibattito su quelle tre parole iniziò in Assemblea costituente e dura ancora oggi. Due sono le opposte tesi messe in campo. Secondo una prima dottrina, tale locuzione si riferisce alle relazioni esterne tra partiti e alla loro attività nella società e nel Parlamento. Contrapposta a questa tesi, vi è però una seconda interpretazione, più diffusa della prima, che vuole che il metodo democratico di cui all'articolo 49 si riferisca alle attività interne dei partiti, al loro funzionamento e alle loro regole interne, nella realizzazione, cioè, del cosiddetto principio di democrazia interna. In questo caso, è necessario un nuovo intervento normativo, una legge che realizzi il principio di democrazia interna per tutti i partiti che concorrono alla politica nazionale e, dunque, alle elezioni politiche nazionali. È in discussione in 1a Commissione qui in Senato il disegno di legge n. 2439 «Norme per favorire la trasparenza e la partecipazione democratica» quale io ed un gruppo di colleghi di molti schieramenti, tutti accomunati dalla militanza politica nel Movimento 5 Stelle in una prima fase, abbiamo presentato l'emendamento 3.1, con il quale vogliamo prendere una posizione netta, chiara e forte nel dibattito, a favore del principio di democrazia interna; posizione supportata anche dalla maggioranza dei costituzionalisti che sono stati auditi in Commissione all'epoca del passaggio alla Camera della legge n. 2439. Su 12 intervenuti su questo tema, infatti, ben otto erano favorevoli a intervenire in qualche forma sul principio di democrazia interna, e di questi quattro erano favorevoli a un intervento molto forte sul tema.

partecipazione e concorso degli iscritti alla determinazione della linea politica; assemblee fisiche dove tale partecipazione e concorso fossero attuate; liste degli iscritti trasparenti; votazioni palesi, salvo i casi previsti dai Regolamenti; garanzia di contraddittorio in caso di provvedimenti disciplinari. Oggi noi siamo fuori da quel partito, perché non c'è nulla di tutto ciò nel Movimento 5 Stelle, e i nostri tentativi di cambiare le cose dall'interno sono falliti. Ora ci stanno pensando i tribunali, a cui si sono rivolti alcuni degli espulsi da quel partito, ad esempio quelli di Napoli e di Genova, che stanno facendo carta straccia delle ballerine e farlocche regole che si sono date al loro interno. Ma noi siamo andati oltre. Noi firmatari oggi crediamo che un partito che non persegua il principio di democrazia interna tramite una manifestazione pubblica di volontà, un vero e proprio statuto redatto in forma di atto pubblico, contenente elementi di democrazia interna a cui esso si obbliga, rappresenti un pericolo per la partecipazione attiva dei cittadini alla politica; si presti a derive del *leader* di turno non facilmente rendicontabili alla comunità; non soddisfi in ultima analisi l'articolo 49 della Costituzione e, dunque, non possa e non debba partecipare alle elezioni politiche nazionali. È questo il senso dell'emendamento che abbiamo presentato in 1a Commissione del Senato al disegno di legge sulla trasparenza dei partiti politici ed è questo il senso di un identico emendamento ormai defunto - l'emendamento 1.26,

laddove l'Italicum aveva inserito l'obbligatorietà della presentazione dello statuto per tutti i partiti che si presentano alle elezioni, anche se l'assenza di un dispositivo sanzionatorio rendeva di fatto vana tale prescrizione. Si tratta di

Tante, troppe volte la politica ha derubricato e rimandato di affrontare questioni cruciali per il buon andamento democratico delle istituzioni, con effetti e ricadute che hanno colpito al cuore il sentimento di partecipazione dei cittadini alla politica, causandone l'allontanamento. Un esempio per tutti è il conflitto di interessi, una vicenda più che ventennale ancora non conclusa, essendo il già citato disegno di legge fermo in 1a Commissione. Un'altro è appunto quello della trasparenza dei partiti, non meno importante, che questo disegno di legge elettorale, malsano nei contenuti e finanche nelle forme con cui è stato imposto ancora una volta con innumerevoli questioni di fiducia, rinuncia a normare. Incredibile quale *cocktail* micidiale stiamo consegnando al Paese, tramite il combinato disposto di questi grandi assenti: conflitto di interessi, trasparenza nei partiti e questo disegno di legge fintamente proporzionale. di legge in elettorale che - lo abbiamo visto - rinuncia a recepire il principio di democrazia interna dei partiti e, anzi, ne peggiora l'attuazione. Il Parlamento della XVIII legislatura che uscirà da questa legge vedrà dunque, in questi scranni un *mix* di parlamentari burattini nominati, manovrati da capocomici o imprenditori in palese o meno palese conflitto di interesse e incapaci di opporsi a ciò che viene dettato loro dalle rispettive sedi aziendali, con dirigenti che si susseguono per successione dinastica da padre in figlio in perfetta identità con il ricambio aziendale. tutte cose che abbiamo già visto e che stiamo vedendo, di cui voi senatori di maggioranza che approverete questo disegno di legge sarete responsabili e conniventi. Ebbene, rimanga agli atti, signor Presidente,

in una riunione dei Capigruppo il 20 dicembre del 2014, alle ore 5,30 del mattino, solo perché Renzi aveva bisogno del suo *spot* elettorale natalizio, voi mi rispondeste laconicamente "si può fare". Così, pacatamente, con l'avallo dell'allora presidente Napolitano, senza troppo rumore, avete spianato le regole costituzionali e il sacrosanto diritto del Parlamento a legiferare. Ho sentito usare parole terribili in quest'Assemblea che, pronunciate con la perversa naturalezza di cui siete capaci, sembrano normali, innocue, ma non lo sono affatto. Il presidente Grasso ha dato il via alla discussione congiunta su cinque - dico cinque - fiducie sul disegno di legge in materia legge elettorale, un abominio procedurale, privando così il Senato della possibilità di migliorare

la terza carica dello Stato, la presidente Boldrini, si è dimenticata di un voto segreto durante la votazione del Tedeschellum

senza la denuncia di quel servizio pubblico - ahimè - in mano al Governo, gestito da fantocci del calibro di Mario Orfeo e dai suoi fedeli amichetti. Attenzione agli amichetti, Orfeo, perché si fa la fine di Dall'Orto.

mai, mai i muri di quest'Aula hanno assorbito tali concetti antidemocratici come un'unica discussione su cinque questioni di fiducia su una legge elettorale: questo significa non poter rappresentare il popolo sovrano.

uno contro l'altro, tradendovi nella strenua lotta per il mantenimento del potere, pronti a tutto, anche all'ennesima larga intesa, eterno progetto così caro al nostro emerito presidente Napolitano.

All'epoca veri uomini e vere donne sedevano su questi scranni a difendere la democrazia dall'autoritarismo fascista e li hanno fermati. Io credo che sia scorretto appellare voi del PD come fascisti, perché siete molto peggio dei fascisti. È un insulto ai fascisti veri. infatti, arrivavano annunciandosi sulle loro camionette cantando: «Allarmi, allarmi siam fascisti», mentre voi, che vi definite eredi dell'antifsascimo, avete tradito il popolo depistandolo in modo vigliacco. In conclusione, signor Presidente, siamo avviliti oltremodo, ma non ci arrendiamo e qua fuori i cittadini protestano, perché oramai è chiaro cosa sta succedendo. Quando il Presidente Grasso (l'equo arbitro), Zanda e le finte opposizioni come Lega Nord e Forza Italia consumeranno questo scempio democratico solo per scambiare un sacchetto di biglie e qualche parlamentare, barattandolo con il loro voto e con il loro riunite qua fuori lo sanno. Sanno che, nonostante i tecnicismi e le perifrasi che usate, li state privando del voto. E nessuno si meraviglierà quando, uscendo di qua, vi sentiranno cantare: «Allarme, allarme siam piddini, terror dei cittadini e della libertà». *(Applausi

meravigliosa Costituzione democratica e antifascista. E lo dico perché comincio a pensare che avete studiato questo pasticcio pensando che il 4 dicembre scorso fosse passata la schifezza di riforma che era stata approvata con gli stessi metodi con cui state procedendo. Dopo il voto

in versione coerente con la schiforma che sarebbe dovuta diventare operativa. Ho pena nel vedere tutte le Province d'Italia, quelle metropolitane e no, abbandonate, senza più risorse, con l'incertezza persino delle lavoratrici e dei lavoratori.

dovete essere prudenti e corretti, perché i danni di tutto questo li hanno pagati i cittadini. Ma almeno lì avevate la speranza di vincere. invece le furbizie, gli stratagemmi e le falsità smaccate non hanno alcun senso. Dove pensate di andare con questo stile? Anche i fedeli nominati, una volta eletti con queste regole, non avendo vincoli di programma, men che mai degli ideali, potranno muoversi a 360 gradi, visto che magari, come è nelle regole della proposta voti un pacifista e viene eletto un interventista, o viceversa; voti un animalista e viene eletto un cacciatore, o viceversa. State scavando la fossa a quel che resta della credibilità della politica e dei partiti. Non me ne compiaccio; anzi so che, quando questo avviene, si aprono sempre scenari spesso drammatici, soprattutto in situazioni come la nostra, dove grande è la sofferenza della popolazione per la mancanza di lavoro, di sicurezza sociale e ambientale e per la totale incertezza dei diritti.

tra le più abominevoli. Il punto è che siete arrivati a questa forzatura totale e finale perché non vi fidate dei vostri parlamentari. È tutto qui.

entrato in una prerogativa esclusiva del Parlamento. Non sapete cosa significhi mantenere la parola ed essere coerenti. State attenti, perché neanche più i finti sondaggi taroccati, quelli che pagate, vi fanno stare tranquilli. Stiamo leggendo tutti, in questi giorni, che li pagate e non se la sentono più di rappresentarvi come l'Italia del mulino bianco. No, ve lo dicono proprio, e a Nord sarà un disastro. un disastro. Eravate tranquilli dopo l'approvazione della controriforma costituzionale, addirittura tracotanti; venivamo insultati,

Lo sanno anche quei deputati e senatori che votano schifezze del genere. Non di fidate di loro e neanche loro si fidano di voi. Ubbidiscono finché sono costretti. La fiducia nei vostri confronti è finita, e per questo abbiamo scritto sui nostri cartelli "zero fiducia". Lo vedremo il cinque novembre in Sicilia e a Ostia; lo vedremo nelle imminenti elezioni nazionali. Dovete correre perché, dopo il voto della Sicilia, nemmeno imponendo la fiducia potreste garantirvi la disciplina dei senatori. Non vi fidate e così fate come con la Costituzione. Ieri avete commemorato la Rivoluzione d'ottobre; dovevate commemorare la disfatta di Caporetto, perché il Rosatellum è questo per voi. Renzi-Cadorna darà la colpa ai fanti e agli ufficiali, quelli che sono andati a rischiare nelle trincee che avete costruito in quel modo. Lui gira in treno a ispezionare le truppe e gli ufficiali, mandando candidature sicure magari in quei collegi all'estero dove avete fatto l'ennesimo imbroglio, dove potranno andare anche gli imbarazzanti per farli votare come quando si nasconde la polvere sotto il tappeto, per capirci.

Avrete compromesso definitivamente ogni capacità di alleanza; andrà bene se la destra prenderà qualche vostro eletto dopo il voto, se gli servirà una manciata di voti,

E le potevate dare con i nostri voti, tra l'altro. Ma non sarà più così. Altri daranno le carte, le destre daranno le carte e potranno essere assolutamente e altrettanto spregiudicate, perché voi avete fatto strame della Costituzione, quella vigente, delle istituzioni, di qualsiasi regola o diritto. Le destre con questa porcheria

Ci sono partiti dentro che hanno un'impostazione nazionalista e centralista, ma che non si sono fatti problemi a dire di costruire l'alleanza. Buon per loro, ma certo questo non può essere la sinistra. Leggo che Renzi farà la campagna sul voto utile. Ma, allora, è come il famoso giapponese dell'isola

Dopo la Sicilia e Ostia, dove non avete matematicamente alcuna possibilità di essere competitivi, il voto utile alla sinistra non può certo guardare al Partito Democratico che, insieme a un pezzo di destra, andrà bene se arriverà terzo tra i contendenti. Gli andrà bene se arriverà terzo. E allora sì che c'è da fare la battaglia per il voto utile a sinistra. Ognuno parli all'elettorato che intende rappresentare in termini di interessi collettivi, di stare dalla parte del mondo del lavoro, dei giovani che non lo hanno, degli anziani per i quali,

E portate i deputati e i senatori come agnelli sacrificali. Con diversi di voi c'era una conoscenza e una stima già da prima. In questi cinque anni ho ed è aumentata la mia stima nei confronti vostri, nei confronti di molti senatori e senatrici, persone che ho conosciuto, capaci e preparate. Non ho problemi ad affermarlo. Per questo concludo dicendo: fermatevi veramente. Altrimenti, vi auguro buona fortuna.

Peraltro, pone la fiducia su questa legge elettorale che è una truffa ai danni dei cittadini e del Paese. Truffa, probabilmente, è il termine che ho sentito maggiormente citare durante questa discussione in Parlamento: legge truffa! Ebbene, io a questo abuso rispondo con le parole di Bertolt Brecht: «Quando l'ingiustizia diventa legge, la resistenza diventa un dovere». *(Applausi dal trio Renzi-Berlsuconi-Verdini al trio Renzi-Berlusconi-Salvini, ma il risultato è esattamente lo stesso. Questo disegno di legge ha uno scopo che è duplice: da una parte, danneggiare la prima forza politica del Paese e mettere in sicurezza il vostro sistema di Governo e di finta opposizione. Avete fatto una legge elettorale incostituzionale, deliberatamente, per rendere più difficile il cambiamento del Paese. Togliete ai cittadini il diritto di scegliere i propri parlamentari, con la falsificazione e la manipolazione del loro voto. Questa è una legge truffa, che illude il cittadino di poter eleggere un proprio rappresentante che può facilmente identificare nel collegio uninominale. Ma, grazie ad artifizi e raggiri, quello stesso cittadino contribuirà invece ad eleggerne altri, non voluti, o addirittura appartenenti a un partito diverso. Verranno eletti nominati dalle segreterie di partito, selezionati in base alla loro attitudine all'obbedienza. Questi parlamentari risponderanno dunque non ai cittadini, ma a chi li ha nominati, e cioè alle segreterie, a loro volta - come sappiamo benissimo - rispondono alle *lobby* di turno, come abbiamo visto ampiamente anche in questa legislatura. E il ciclo continua, a tutto danno della democrazia, a danno dei cittadini e a danno del Paese. Questa legge non porterà neanche stabilità al Paese. Secondo i maggiori osservatori e analisti, non darà proprio alcuna possibilità di governare. questo rende di tutta evidenza la necessità, per la formazione di una maggioranza e la nascita di un Governo, di fare una coalizione di coalizioni, o, quantomeno, di una unione incestuosa tra i due principali gruppi avversari, Partito democratico e Forza Italia, avversari ovviamente solo di facciata, solo per il tempo della campagna elettorale. Insomma, il disegno sembra essere fin troppo chiaro: creare un nuovo Governo di conservazione, Renzi-Berlusconi. Ma la sola convergenza tra Partito Democratico e Forza Italia non sarebbe stata sufficiente. C'era bisogno di un "utile idiota" che portasse un ulteriore e necessario contributo di consenso. E prontamente eccolo lì che spunta: si chiama Matteo Salvini. D'altra parte, come già efficacemente ricordato dal collega Endrizzi,

unicamente finalizzate al momento elettorale. Pensate, ad esempio, alla Lega, che, fresca di *referendum* per l'autonomia in Veneto e in Lombardia, già annuncia alleanze con i partiti centralisti, che hanno già bocciato ogni ipotesi di decentramento qui in Parlamento. Insomma, l'unico scopo è quello di incassare qualche seggio in più, senza alcuna condivisione di un progetto, senza alcuna condivisione di un programma, senza alcuna condivisione di un candidato *Premier*. di legge consentirà, tra l'altro, ad un ex *leader* politico pregiudicato di vedere stampato il proprio nome sulla scheda elettorale, nonostante sia stato interdetto dai pubblici uffici, nonostante per la legge italiana non si possa candidare o ricoprire un ruolo di Governo.

è per caso lo stesso della P2, dei rapporti con la mafia, delle tangenti, della compravendita dei giudici, della compravendita di parlamentari, dei falsi in bilancio, delle frodi fiscali, dei conflitti di interesse, delle leggi *ad personam*? No, non può essere lui, non è possibile. *(M5S)*. Non è possibile. Eppure, per danneggiare il Movimento 5 Stelle state superando ogni peggiore immaginazione, state facendo ripiombare il Paese che amiamo e che necessita di entrare nel futuro, nel suo peggior passato. Concludo, Presidente. Insomma, state umiliando milioni di cittadini onesti e credete di poterla fare franca. Credo che vi stiate sbagliando, perché state sottovalutando l'intelligenza dei cittadini, state sottovalutando la volontà, il desiderio di milioni di persone di partecipare alla vita politica del Paese, milioni di persone che si sentono oggi defraudate di uno dei loro diritti più importanti, quello di decidere per chi votare. Credete che gli italiani si bevano di tutto. Io credo che vi sbagliate. Questa legge sarà un *boomerang* che vi rivolgerà contro perché non si può arrestare un moto di cambiamento che è già maturo nel Paese. I cittadini stanno sempre più acquisendo la consapevolezza del fatto che il vostro "Imbrogliellum" è solo una truffa e da truffati se ne ricorderanno alle prossime elezioni.

che un sistema elettorale possa stravolgere una volontà popolare. Penso che bisogna stare attenti

che questa è una legislatura iniziata all'insegna della dubbia legittimità del Parlamento in ragione della legge elettorale utilizzata per costituirlo. Il Porcellum è stato sottoposto all'esame della Corte costituzionale, la quale ha individuato nel Porcellum difetti costituzionalmente rilevanti tanto da intervenire con una propria sentenza a ridurne la capacità di intervento. Quindi un obbligo avevamo, lo disse la stessa Corte costituzionale nel licenziare la sentenza: avevamo l'obbligo di affrontare il problema del sistema elettorale e di restituire ai cittadini una legge elettorale legittima sotto il profilo costituzionale. Abbiamo iniziato questa legislatura con grande difficoltà e prendiamo atto di un altro elemento: nessuno schieramento politico, nessuna coalizione omogenea aveva vinto le elezioni. Avevamo quindi una legge elettorale incostituzionale e una inesistente maggioranza politica, venuta fuori dal risultato elettorale.

nel Parlamento italiano, con la maggioranza certa all'interno della Camera dei deputati. Non ho partecipato, anzi, ho fatto opposizione per diversi anni, ma ricordo quei giorni, quei mesi e gli sforzi fatti da tutti per avviare un processo di riforma costituzionale che ricomprendesse anche la legge elettorale. Ne Ne deriva quindi una cosa: noi da questo Parlamento non potevamo andare via senza aver compiuto il nostro primo dovere, cioè quello di restituire ai cittadini italiani una legge elettorale costituzionalmente garantita. Questo lavoro è stato per una certa fase accompagnato anche da una volontà riformatrice più ampia.

e per mesi e per anni ne abbiamo discusso in questo Parlamento, anche in maniera molto accesa. Tanto abbiamo discusso che siamo andati con una riforma costituzionale approvata dal Parlamento, a larghissima maggioranza, ad un confronto con il Paese attraverso un *referendum* confermativo. Io ho votato no

che secondo me mortificava le autonomie esaltando un centralismo o neocentralismo dello Stato nazionale, dello Stato nazionale, era accompagnato da una legge elettorale conforme a quel tipo di riforma. Per cui ci siamo ritrovati una legge elettorale approvata, forse costituzionalmente valida ma inefficace rispetto ad un altro sistema costituzionale, che era quello dell'inizio della legislatura, perché quel provvedimento rispecchiava esigenze che erano state espresse nella riforma costituzionale approvata dal Parlamento e poi bocciata dal successivo *referendum* confermativo. Quindi

non abbiamo l'ambizione di rappresentare movimenti politici e per noi vale il ragionamento che facciamo da parlamentari, assumendoci la responsabilità di quello che facciamo - oggi vale votare questa proposta di legge elettorale, perché così adempiamo ad un dovere che abbiamo ritenuto di assumerci quando abbiamo votato la fiducia al Governo Gentiloni Noi, io e il collega Dario Stefano per primo, per la prima volta in questa legislatura, abbiamo votato la fiducia ad un Governo. E lo abbiamo fatto per dare una risposta a delle preoccupazioni esistenti: preoccupazione della messa in sicurezza dei conti, perché questo è un Paese che esce dalla crisi, che è stata sofferta dai cittadini e non dai parlamentari, e, e, uscendo dalla crisi, non bisogna mai buttare il lavoro fatto, ma occorre conservarlo e partire da quello, per farne uno migliore;

politica continua a sviluppare, qualcuno pensa di esserne danneggiato e qualcun altro pensa di esserne favorito. La realtà è che, molte volte, quelli che pensano di essere favoriti poi finiranno per essere danneggiati e quelli che pensano di essere danneggiati forse

non mette in discussione nessuna delle difficoltà che intravediamo, anche nel testo che verrà approvato. Ce ne sono, anche di natura tecnica, anche nell'assegnazione dei seggi e ci sarà una discussione anche giuridica oltre che nelle sedi proprie, per capire come verranno assegnati i parlamentari alle diverse coalizioni e forze politiche. Voglio

consente la formazione di coalizioni omogenee, consente garanzie per ciò che riguarda la parità di genere e consente, soprattutto, l'armonizzazione dei sistemi elettivi di Camera e Senato, che era una delle

frutto di due sentenze della Consulta e della bocciatura delle riforme costituzionali. Per effetto di queste due cause, l'Italia non dispone oggi di una legge elettorale coerente per i due rami del Parlamento e non dispone neppure di una legge comunque operativa, perché se vivesse il Consultellum sarebbe necessario un intervento normativo di armonizzazione tra Camera e Senato. Era dunque necessario porre rimedio, con una legge che in primo luogo rispettasse il dettato delle due sentenze della Corte e che mettesse d'accordo una maggioranza parlamentare, la più ampia possibile, anche perché sarebbe stato almeno sconveniente per il legislatore, dal punto di vista istituzionale, non tentare di rispondere ai ripetuti appelli del Capo dello Stato affinché si varasse una legge elettorale condivisa. Dopo il tentativo fallito del giugno scorso, quando una maggioranza bulgara non è riuscita a portare a casa il risultato, fermandosi al primo voto segreto, rischiare un fallimento anche oggi, alle porte dello scioglimento della legislatura e con una delicatissima legge di bilancio ancora tutta da scrivere, sarebbe stato troppo pericoloso. Pericoloso per la tenuta democratica di un Paese Pericoloso per la tenuta democratica di un Paese non è certo approvare una legge elettorale col voto di fiducia; lo sarebbe, invece, arrivare a pochi mesi delle elezioni avendo come sistema elettorale vigente "due residuati bellici" come li ha definiti il Presidente emerito della Corte costituzionale, Valerio Onida. Due residuati bellici dannosi e inutilizzabili. Inutilizzabili, perché a quelle leggi mancano del tutto le norme per consentire l'espressione del voto di preferenza al Senato e, sempre al Senato, non si sa se potrebbero formarsi coalizioni

Un *caos* apparentemente calmo che somiglia molto alla quiete che precede la tempesta. E dunque ricorrere al voto di fiducia per prevenire la tempesta di un prossimo Parlamento certamente ingovernabile non va considerato come un attacco alla democrazia, semmai come un atto di responsabilità. Una responsabilità politica a cui non ci sottrarremo, in coerenza con quanto abbiamo sempre fatto nel corso di tutta questa legislatura - senza mai chiedere nulla in cambio - anche perché questa legge abbiamo contribuito a scriverla alla Camera e lo facciamo ancora oggi allo scopo di garantirne l'approvazione in tempi rapidi e senza rischi inutili. D'altronde, la storia di questo Parlamento è ricca di provvedimenti cruciali caduti sotto i colpi dei franchi tiratori. Agguati mossi nell'ombra, com'è avvenuto alla Camera qualche mese fa, all'insegna del tanto peggio, tanto meglio. Voglio poi ricordare cosa ci ha chiesto la Consulta con le sue sentenze del 2013 e del 2017: una legge con liste corte di candidati o collegi uninominali, una legge uniforme per le due Camere, una legge con un automatismo per l'opzione del plurieletto: tutte caratteristiche proprie del Rosatellum. C'erano altri punti sollevati dalla Corte, aspetti della legge che sarebbero stati considerati legittimi a determinate condizioni. Uno fra tutti è il premio di maggioranza. Noi avevamo chiesto una legge che fosse almeno in parte maggioritaria, presentando un testo con il 50 per cento di collegi e il 50 per cento di listini proporzionali. Abbiamo poi votato sì alla Camera al Rosatellum nella sua prima versione, ci siamo opposti senza sbraitare al sistema proporzionale tedesco e oggi non possiamo che essere quota fosse stata più alta, con un premio o con un numero maggiore di collegi. Oggi diciamo che va bene così, anche se resta penalizzato il valore della governabilità, valore che non può essere sacrificato sull'altare della rappresentanza a ogni costo. Rappresentanza senza correttivi maggioritari significa spesso ingovernabilità; si pensi, per un attimo, alla Germania di Weimar e alla Francia della quarta Repubblica, senza dimenticare la nostra prima Repubblica con i suoi cinquanta I sistemi maggioritari o almeno misti sembrano meglio rispondere alle esigenze della modernità, dando la possibilità di avere un vincitore all'esito delle elezioni e stabilità ai Governi. Solo negli ultimi anni, le grandi nazioni europee sull'orlo di crisi istituzionali a causa del proporzionale sono state molte: il Belgio per diciotto mesi non ha avuto Esecutivo; la Spagna e la Grecia sono andate alle urne due volte in dodici mesi e adesso la Germania probabilmente sarà costretta a una coalizione che andrà dai liberali ai verdi, passando per i democristiani. Dunque noi abbiamo prima di tutto il dovere di dotare il Paese di un sistema il più possibile efficiente e coerente, rispondendo, come ho già detto, ai ripetuti appelli rivolti dal Presidente della Repubblica. Questa legge almeno una sua coerenza tra Camera e Senato ce l'ha; quanto alla sua efficienza, ossia alla possibilità di formare una maggioranza politica omogenea mancando un significativo premio di maggioranza, i dubbi sono legittimi: dipenderà dalla campagna elettorale e dall'offerta politica che sapranno presentare le coalizioni. Ma è chiaro che in un sistema tripolare l'unica vera garanzia di governabilità la darebbe il ballottaggio, che nell'Italicum era previsto e che la Consulta ha di fatto reso irrealizzabile. In questa situazione, che senso ha demonizzare le coalizioni, la cui introduzione è costata al Rosatellum addirittura la definizione di «legge criminale»? Qui, questo autorevole critico ha dimostrato di avere davvero la memoria corta. Ricordo, infatti, che l'Italicum era stato definito da molti come una legge eversiva perché avrebbe favorito l'avvento Grazie che le coalizioni esistono già nelle leggi per i Comuni e per le Regioni (leggi evidentemente criminali anche quelle…), e non mi sembra che qualcuno le abbia tacciate di antidemocraticità. Coalizioni, peraltro, che sarebbero ricomparse anche con il Consultellum, perché ancora esistenti per il Senato. Il vero problema di cui si può e si deve discutere, come ho già accennato, è se questa legge risponda al requisito della governabilità. Da questo punto di vista, il Rosatellum ha un correttivo maggioritario modesto, ma sinceramente non si poteva fare di più, visti i paletti rigidi posti dalla Consulta sul problema della rappresentanza. Tuttavia, poiché nei 232 collegi vince chi arriva primo, è possibile che una coalizione di liste o una lista singola se ne aggiudichino una gran parte. La cancelliera Merkel, lo scorso settembre, con il 33 per cento dei voti ha conquistato il 77 per cento dei collegi uninominali. Anche in presenza di un distacco minimo fra primo e secondo, dunque, può verificarsi una vittoria netta nei collegi. Dipenderà dalla campagna elettorale, che una quota di voti li sposta sempre, dall'organizzazione dell'offerta politica e ovviamente dalle scelte degli elettori. Cosa che normalmente accade quando siamo in presenza di leggi elettorali democratiche, come a tutti gli effetti è il Rosatellum. Si tratta di una legge non certo perfetta, ma parlare di colpo di Stato è veramente ridicolo, oltre che pericoloso.

Ci hanno risparmiato la fiducia soltanto su uno degli articoli della legge, l'articolo 5, che è quello dell'invarianza finanziaria. Per il resto, tutta la legge, l'intero l'articolato è stato sottoposti al voto di fiducia. La prima domanda che ci si pone e che si dovrebbe porre chiunque è: come mai il voto di fiducia? Su questo abbiamo due interpretazioni possibili,

L'altra possibilità è che qualcuno lo abbia chiesto e cioè che prevalga un'altra versione, che pure è stata offerta all'opinione pubblica, secondo cui il Governo non ha posto

la fiducia con dichiarazioni programmatiche che oggi vengono smentite. Ricordo le frasi - e le voglio leggere - del «Lascio alla dialettica tra le forze politiche il dibattito sulla durata del nuovo Governo. Per quanto ci riguarda, vale la Costituzione: il Governo dura quando ha la fiducia

l'altra attività - «alla nostra agenda, prenderà corpo il confronto tra le forze parlamentari sulla legge elettorale e sulla necessaria armonizzazione delle norme tra Camera e Senato. È un confronto nel quale il Governo - voglio ribadirlo, come ho avuto occasione già di dire negli incontri con le diverse delegazioni non sarà l'attore protagonista. Spetta a voi, onorevoli colleghi, la responsabilità di promuovere e trovare intese efficaci. Certo, il Governo non starà alla finestra, cercherà di accompagnare, di facilitare e anche di sollecitare questo confronto. La sollecitudine non deriva dalle valutazioni sulla durata dell'Esecutivo, deriva dalla consapevolezza Ebbene, da queste dichiarazioni programmatiche al voto di fiducia vi è uno scarto logico che non è facile da capire, soprattutto se si considera Grazie a seguire una strada di collaborazione e di accompagnamento, ma non ad avere, come ha oggi, apponendo la fiducia, un ruolo da protagonista. Forse Gentiloni Silveri è già consapevole che la maggioranza di allora non è la maggioranza di oggi,

sta seguendo forse le indicazioni di una minoranza che lo tiene al Governo? Sono tutte considerazioni che verificheremo sul campo. Voglio sul punto soltanto richiamare un'affermazione del capogruppo del PD Zanda, che - è evidente - da esperto stratega di dinamiche parlamentari sa bene cosa succederà in quest'Aula. Ebbene Zanda dice che i cinque voti di fiducia chiesti al Senato dal Governo per l'approvazione della riforma elettorale sono un elemento tecnico.

del fatto che il Governo, per avere numeri sufficienti per far passare questa legge elettorale, ha bisogno di appoggi. Non solo, probabilmente, dell'appoggio di chi si allontanerà e dell'appoggio che abbiamo già visto (in questa triste vicenda abbiamo una certa esperienza), ma anche di appoggi concreti visibili,

e chi osserva le dinamiche parlamentari con responsabilità ben più alte dovranno prendere atto che la maggioranza che ha dato fiducia al Governo Gentiloni Silveri nel dicembre 2016 non c'è più e che, se c'è una nuova maggioranza, bisogna procedere con una crisi di Governo. Non conosco altre strade, almeno se le regole del diritto parlamentare, che molti di voi qui dentro potrebbero sicuramente insegnare a me, sono ancora valide. E adesso vorrei fare delle osservazioni

più spesso citata come governabilità, la stabilità del Governo. Ebbene, credo che questo valore, che è sicuramente di rilevanza costituzionale, venga citato abbastanza a sproposito. Ricordo a tutti che in quella sentenza la Corte ne parla Corte ne parla perché sta valutando il premio di maggioranza - che poi dichiarerà incostituzionale - e, per spiegare i limiti che un legislatore ha, sostiene che i valori costituzionali e innanzitutto gli articoli 1, 3 e 48 secondo comma, della Costituzione,

possono essere compressi. I sistemi elettorali spesso comportano delle compromissioni, ma compromissioni serie, di una certa rilevanza possono essere giustificate soltanto dal conseguimento di obiettivi di rilevanza costituzionale come ad esempio, nello specifico, la stabilità

dovrebbe garantire il valore della rappresentatività. Non stiamo dunque introducendo distorsioni per garantire governabilità, ma stiamo

prendono parte? Dove sono i membri di Forza Italia? Perché le coalizioni farlocche di cui stiamo parlando, con programmi diversi e con *leader* diversi, non servono a Renzi, ma servono a scrivere i nomi di Berlusconi, Salvini e Meloni, per unire in coalizioni che si divideranno con programmi diversi il giorno dopo, servono a garantire quello che dice Salvini: sarà il *leader* che avrà più voti. Ebbene, non ci avete consentito di discutere nel merito e non avete consentito a questa Assemblea di discutere nel merito neanche su elementi

È incredibile che con il voto di fiducia si ottenga che la Commissione che dovrà disegnare i collegi sarà di nomina esclusivamente e che non ci sarà nessuna partecipazione alla nomina del Presidente del Senato, né della Presidente della Camera, cioè di organi e soggetti imparziali.

Signor Presidente, la ringrazio in modo particolare per aver voluto considerare le mie difficoltà personali, consentendomi di prendere la parola da seduto a questo banco. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, il così controverso *iter* della nuova legge elettorale ha portato in primo piano esigenze e ragioni non facilmente componibili tra loro, da considerare tuttavia non solo in riferimento ad una pur rilevante, drammatica contingenza come quella di cui parliamo. Da un lato è emersa con forza un'esigenza da tempo presente nell'esperienza e nell'evoluzione della vita pubblica, non soltanto in Italia: parlo della capacità di decisione del sistema democratico di fronte a cambiamenti epocali che richiedono risposte tempestive e incisive da parte delle *leadership* di Governo. questione che si acuisce quando si tratti di approvare provvedimenti volti a risolvere problemi d'innovazione e cambiamento da troppo tempo sterilmente dibattuti e rimasti irrisolti. Dall'altro lato - e qui ho ritenuto e ritengo di dover porre un mio personale forte accento - emergono le ragioni dell'equilibrio tra le istituzioni, i poteri e i ruoli propri di ciascuna di esse nell'ambito dei singoli ordinamenti costituzionali e in coerenza con l'assetto europeo. Vorrei che almeno nel prossimo futuro, in diverse condizioni, si potesse tra le forze politiche in seno al Parlamento discutere di tali questioni come questioni di interesse generale e di comune responsabilità politico-istituzionale. Ma si può far valere l'indubbia esigenza di una capacità di decisione rapida da parte del Parlamento fino a comprimerne drasticamente ruolo e diritti, sia della istituzione, sia dei singoli deputati e senatori? L'interrogativo è sorto in concreto nelle ultime settimane con la decisione del Governo di apporre la fiducia sulle parti sostanziali del testo, prima che si aprisse in Aula alla Camera il confronto sugli emendamenti all'articolo 1. Ma mi domando, al di là delle opposte posizioni espresse notoriamente a quel proposito dalle forze politico-parlamentari: esiste o no un dilemma di carattere generale da discutere insieme e in prospettiva? Il dilemma non è fiducia o non fiducia, anche perché non è mai stata affrontata neppure dinanzi alla Corte costituzionale un'obiezione di incostituzionalità della fiducia. C'è però stato nell'esperienza italiana ricorso alla fiducia in occasioni e in modalità molto diverse tra loro. loro. Quali forzature può implicare e produrre il ricorso a una fiducia che sancisca la totale inemendabilità di una proposta di legge estremamente impegnativa e delicata? È questo il punto che ho sollevato con le riserve e posizioni espresse nella vicenda concreta che si sta concludendo in sede parlamentare. È questo che mi premeva, assai più che auspicare una specifica modifica al testo. In effetti, l'auspicio da parte mia era che si eliminasse l'ultima sopravvivenza della legge Calderoli, promulgata nel 2005.

della clausola relativa all'indicazione, in sede di procedimento elettorale, dei nomi del capo della forza politica e soprattutto del capo della coalizione. Quell'auspicio partiva dall'esperienza da me fatta, come Presidente della Repubblica, degli equivoci che di lì erano scaturiti sul piano degli equilibri costituzionali, adombrando un'elezione diretta del Presidente del Consiglio. Il punto critico era dunque ai miei occhi quello - ripeto - della totale inemendabilità della proposta di nuova legge elettorale. Ora, sia chiaro - non dovrebbe essere necessario ricordarlo - che nessuno più di me poteva auspicare, all'unisono con il presidente Mattarella, l'approvazione più largamente condivisa dal Parlamento di una nuova legge elettorale. Questa per circostanze ben note era diventata urgente, anche se dovremmo essere consapevoli dell'anomalia di troppi, frequenti cambiamenti in Italia di una disciplina, come quella elettorale, che dovrebbe essere (ed è generalmente in Europa) costante per un lungo periodo e non essere modificata alla vigilia di elezioni politiche generali. Siamo sicuri che quella ora in votazione possa reggere a lungo, che abbia un fondamento sufficientemente solido da proiettarsi in un orizzonte di ragionevole durata? Ben prima di essere eletto Presidente e poi nell'esercizio del mio mandato, avevo sollecitato e poi assunto come obbiettivo fondamentale nell'interesse del Paese l'adozione sia di una nuova legge elettorale, sia della riforma della seconda parte della Costituzione, ma mi trovai dinanzi a un nulla di fatto in tutta la legislatura 2008-2013, nonostante la formale condivisione di quegli obbiettivi da parte di partiti di entrambi gli schieramenti e a dispetto di promesse da essi fatte e non mantenute. Nel merito, ho apprezzato la scelta di fondare la nuova legge elettorale su un *mix* di proporzionale e maggioritario, nella scia della legge Mattarella del 1993, dalla quale però sarebbe stato coerente mutuare anche la netta distinzione tra le candidature nei collegi e quelle nelle liste dei partiti *(Applausi davvero non un semplice tecnicismo, come si è detto. Infine, singolare e sommamente improprio ho trovato il far pesare sul Presidente del Consiglio la responsabilità di una fiducia che garantisse la intangibilità della proposta in quanto condivisa da un gran numero di partiti. Il presidente Gentiloni Silveri, sottoposto a forti pressioni, ha dovuto aderire - e me ne rammarico - a quella convergente richiesta, proveniente peraltro da quanti avrebbero potuto chiedere il ricorso alla fiducia non già su tutte le parti sostanziali della legge, ma su punti considerati determinanti, che non ebbero la lucidità e il coraggio di fare. In definitiva, ho compreso la difficoltà in cui si è trovato un Presidente del Consiglio che ho stimato e stimo per il modo in cui ha guidato e guida il Paese, rafforzando la posizione dell'Italia come interlocutore valido sul piano europeo e internazionale. Altro tema che si è presentato in rapporto a questa vicenda e resta, onorevoli colleghi, per tutti noi da meditare è quello del come contrastare forme di ostruzionismo dilatorio o paralizzante in Parlamento. Il tema è stato oggetto di una lunga storia in Italia, a partire da efficaci interventi già negli anni della presidenza Iotti alla Camera. In verità, su quella strada si sarebbe potuti andare più avanti, se non fossero ad esempio rimasti sempre nel cassetto progetti di riforma dei Regolamenti parlamentari. Detto ciò, è corretto sostenere che oggi una linea antiostruzionistica può affidarsi solo a mezzi estremi come il vanificare ogni ricorso all'istituto del voto segreto e il negare ogni libero confronto emendativo? E ciò a prezzo di qualunque costrizione di diritti e di ruolo del Parlamento e dei singoli parlamentari? Converrebbe, Converrebbe, onorevoli colleghi, pensarci bene tutti. Si sa qual è stata la mia identificazione, potrei dire per un'intera vita, con la causa del fondamento parlamentare nella nostra democrazia costituzionale. Ma è stata per me essenziale e tale resta la necessità in pari tempo di misure e comportamenti miranti a una maggiore funzionalità, efficienza produttività nello svolgimento dei lavori parlamentari, anche attraverso lo sveltimento e la prevedibilità dei tempi dell'esame di ogni provvedimento nelle Camere, senza che il Parlamento stesso esorbiti peraltro dalle sue funzioni. Tutto questo è essenziale anche per contrastare i rigurgiti di una campagna antiparlamentaristica che conta tristi precedenti storici in Italia. Signor Presidente, onorevoli colleghi, al punto in cui siamo occorre guardare avanti, innanzitutto alla necessità di salvaguardare due beni vitali per l'Italia: la stabilità di Governo e lo sviluppo di una funzione assertiva e costruttiva del nostro Paese nel processo di integrazione e unità dell'Europa, cui è legato fondamentalmente il nostro comune destino. Più in generale, vorrei richiamare il modo in cui, nell'estate 2011, cercai di trarre le principali lezioni dall'esperienza del centocinquantenario dell'Unità d'Italia. Lo feci parlando a una vasta assemblea di giovani, nel contesto indipendente del *meeting* di Rimini. Mi impegnai lì in un discorso di ampia prospettiva, oltre i tradizionali steccati politici: occorre mirare, dissi, a un grande sforzo collettivo - nato da un comune esame di coscienza - come quello da cui scaturì, dopo la liberazione dal nazifascismo, la ricostruzione democratica, materiale e morale del nostro Paese, cui - voglio ricordarlo - si accompagnò la salvaguardia dell'unità nazionale, messa in questione da impulsi separatisti e da pressioni dei Paesi confinanti.

del nostro tempo a rappresentare la molla per procedere in quella direzione. Si richiede però più obbiettività nelle analisi e nei giudizi, più apertura e meno insofferenza verso le voci critiche e le opinioni altrui. C'è - diciamolo chiaramente - da risalire la china della sedimentazione in questi decenni, nella sfera della politica, di chiusure, di faziosità, di derive verso meri scontri di potere e anche di personalismi dilaganti come non mai in seno a ogni parte. La prospettiva - ribadisco oggi - non può essere che una: un nuovo senso di comune responsabilità, al di là delle alterne vicende della competizione politico-democratica e quindi della collocazione, in ciascun periodo, dei singoli partiti in maggioranza o all'opposizione. Solo così possiamo fare i conti con la vera e propria crisi di sistema che stiamo vivendo in Italia e altrove. Come ha di recente scritto uno dei nostri maggiori studiosi e analisti dei fondamenti e dei percorsi della politica, ci ci dibattiamo in quello che è perfino in qualche modo un "nuovo caos", di fronte a fenomeni come il prevalere delle "particolarità dei sentimenti e delle passioni", di psicosi, di allarme e paura e di istinti di autodifesa: quasi che - secondo le parole dello studioso - "la democrazia stesse perdendo la ragione", perdendo così irrimediabilmente se stessa. Dunque è il momento, io ritengo e vorrei che su ciò consentissimo, di sollevare lo sguardo dallo scontro quotidiano, dalle sue angustie e dalle sue nevrosi di "fine legislatura". In questo spirito preannuncio, con tutte le problematicità e le riserve che ho cercato di motivare, la fiducia al Governo Gentiloni Silveri per salvaguardare il valore della stabilità,

prerogative attribuitegli dalla Costituzione e dalle leggi. Grazie per l'attenzione.

questa legislatura è iniziata male e si accinge a chiudere nel peggiore dei modi. Chiudiamo, cioè, la legislatura con una nuova proposta di legge elettorale. Forse è meglio ripeterlo, perché credo che ai più il fatto appaia del tutto naturale. Chiudiamo la legislatura votando una nuova legge elettorale, cioè, mi ripeto, a pochi mesi dalla scadenza elettorale, oppure - provo a trovare anche un diverso punto di vista - a pochi mesi dalla scadenza del mandato parlamentare, questo Parlamento licenzierà le nuove regole per le prossime elezioni politiche. Tutto ciò sulle note di quella insostenibile leggerezza dell'essere che ha animato la politica di questi ultimi vent'anni e che si è magicamente trasferita su quel Matteo Renzi che credo passerà alla storia,

sono certo che stiamo commettendo una leggerezza che peserà come un macigno sul futuro delle istituzioni democratiche. Noi statuiamo, cioè, che ogni e qualsiasi futura coalizione o partito potrà, *in limine* del proprio mandato, farsi la legge elettorale che più gli aggrada. E lo facciamo con una sufficienza tale che il voto di fiducia appare quasi l'infiocchettamento naturale di cotanta arroganza. Lo capisci nel candore con il quale il senatore Zanda, davanti alle telecamere sostiene la correttezza di tale scelta. E allora la mente corre ai buoni studi passati e torni allo spirito che aveva animato le scelte dei senatori Romani, quello spirito che faceva ritenere l'età sinonimo di saggezza. Ecco, io sono qui a chiedermi: dove è finita la saggezza degli anziani? Dove è il senso dello Stato? Dove è la cura delle istituzioni e - vivaddio - dove è finito il buon senso? E ancora, dove è finito il dibattito parlamentare? Raccontare questa legislatura sarebbe come raccontare con quanta arroganza e tracotanza si è fatto strame di norme, leggi, regolamenti parlamentari, consuetudini e buon senso. Una legislatura passata sotto il maglio del voto di fiducia. Ma per un attimo vogliamo interrogarci e chiederci cosa sia il voto di fiducia? Nella dialettica parlamentare il voto di fiducia è il momento politico più alto: una corale assunzione di responsabilità rispetto ad un progetto, ad un programma ad una visione. Purtroppo, constatiamo che nella realtà odierna questo strumento è stato svilito ad un dozzinale mezzuccio attraverso il quale qualche potente di turno impone la legge del più forte, rappresentando un monocameralismo fuori da tutte le garanzie costituzionali. E il Senato diventa un orpello dentro il quale il confronto viene seppellito e il dissenso silenziato e disinnescato con il voto di fiducia. Ho il piacere di intervenire dopo il presidente Napolitano, ma non so se guardare con sospetto o con la bonomia che esige il rispetto per l'età a questa sua tardiva resipiscenza. Dello scempio delle regole parlamentari il presidente Napolitano, infatti, è stato - a mio avviso - uno spettatore distratto. Durante il suo secondo mandato un suo messaggio alle Camere sulla decretazione d'urgenza

E anche molti di quelli che quel risultato hanno determinato assistono oggi all'usurpazione delle nostre prerogative parlamentari in un religioso silenzio. Ma come si fa a licenziare un disegno di legge di riforma elettorale (lo ripeto, una legge di riforma elettorale) senza dibattito parlamentare, senza che i senatori possano discutere, verificare ed emendare? Abbiamo dedicato molto più tempo al provvedimento su Sappada, signor Presidente, o alla commemorazione del bicentenario di Bellini (neanche ricordo di chi si Ecco, questo è uno dei tanti precedenti disastrosi che questa legislatura ha collezionato. Per la prima volta nella storia repubblicana il Senato viene sollevato dalle sue funzioni sulla proposta di una legge di riforma del sistema elettorale. Assisto attonito ad una deriva che, peraltro, denuncio da tempo, cioè la sistematica esautorazione della funzione legislativa da parte del potere esecutivo sul potere legislativo. Le leggi le fa e le deve fare il Parlamento, come diretta emanazione del popolo. Non può e non deve farle il Governo o un Capo di Governo. Dobbiamo porre un argine a questo tentativo subdolo di insinuare un uomo solo al comando, o un manipolo di pochi, a dispetto di un sistema che continua a professarsi democratico. Non dobbiamo più permettere che ci vengano sottratti spazi di democrazia. Signor Presidente non conosco, non avendone avuto il modo, questa legge elettorale. E le consegno, signor Presidente, questa come una mia denuncia, perché qualcuno fa menzione di di un passato che è completamente diverso da quello che stiamo vivendo. Infatti, se qualcuno guardasse bene alla storia della legge truffa, ricorderebbe che vi sono stati dei passaggi parlamentari estremamente significativi.

signor Presidente, siccome lei dovrebbe e deve difendere le nostre prerogative, consegno a lei questa mia denuncia. Quindi, non conoscendola non potrò votare questa riforma questa riforma elettorale né tantomeno potrò votare la fiducia o le fiducie che sono state richieste perché, citando un autorevole autore toscano, «'l modo ancor m'offende».

tre voti di fiducia alla Camera e cinque in Senato: è evidente che il Governo Gentiloni Silveri e la maggioranza che lo sostiene devono avere davvero a cuore questo disegno di legge elettorale, detto Rosatellum. Eppure, tutti ricorderete come due anni fa la stessa maggioranza e un Governo del quale il presidente Gentiloni Silveri si considera l'erede, il continuatore, abbiano, sempre con la fiducia, fatto votare una legge elettorale che era assolutamente l'opposto di quella oggi in discussione. L'Italicum, infatti, escludeva le coalizioni, considerandole di competizione interna e dunque di ingovernabilità. Il Rosatellum le ripesca e le libera dalla necessità di formare un Governo comune; quindi, le fa diventare un semplice strumento per ramazzare voti. L'Italicum aveva un premio di maggioranza obbligatorio che scattava sempre al secondo turno, e Renzi disse che la sera stessa si sarebbe Il Rosatellum non ha il premio di maggioranza e probabilmente renderà più difficile formare un Governo dopo il voto, perché le coalizioni elettorali che si sono formate verosimilmente si dovranno rompere per costruire diversi equilibri. Uno studioso delle nostre vicende istituzionali si chiederebbe com'è possibile questa mutevolezza dell'orientamento della maggioranza, accompagnata, però, da una comune, continua insistenza e passione per il voto di fiducia. Come nei gialli, la risposta è semplice: in questo caso, i secondi e i terzi si sono messi d'accordo per togliere la vittoria ai primi. Tutti sapete, infatti - fuori di qui se ne parla ogni giorno - che i sondaggi dicono che, se si votasse oggi,

se passa una legge che prevede coalizioni senza l'obbligo del programma, per Forza Italia, per la Lega Nord e per il Meloni, sarà possibile mettersi insieme senza bisogno di costruire un programma di Governo e di indicare un *Premier*. Allora, probabilmente - dicono i sondaggi - la prima forza non sarebbe più

e far passare anche all'estero questa versione dei fatti? Per capirlo dobbiamo ritornare a quello che è successo alcune settimane fa. Il Partito Democratico aveva chiuso, con il Movimento 5 Stelle e con Forza Italia, un accordo per una diversa legge elettorale. Poi, però, davanti a un emendamento tutto sommato marginale, che metteva in questione l'alleanza con una forza autonomista, ma sostanzialmente marginale, è stato il Partito Democratico a ritirare di legge. Perché? Molto semplice: si sono resi conto al Nazareno che lo sbarramento che quella legge prevedeva avrebbe favorito il formarsi di una lista unica non solo tra Sinistra Italiana 1-Movimento democratico e progressista, ma anche, forse, addirittura con Campo Progressista. Allora si ferma tutto, si torna indietro e si creano quelle coalizioni che fino a ieri costituivano la ragione di ingovernabilità perché con esse si possono fare due operazioni una parte, giocando sul voto utile e presentando lo spauracchio della destra, che si è favorita con la legge elettorale, si può dire «venite da noi», senza alcun impegno programmatico e senza rivedere nulla delle scelte fatte durante la legislatura, ma soltanto accomodandovi con

per la Sardegna, sostenuta da un sindaco *ex* arancione; ci può essere una lista Verdi, un po' radicali, con una tintura di Ulivo.

costruire una maggioranza di Governo sarebbe più difficile che se ci fosse stata una pura legge proporzionale. Tutto questo sarebbe però da parte mia non generoso. Guardando infatti ciò che è avvenuto in questa legislatura, devo riconoscere che non c'è soltanto uno spirito tattico immediato nel processo che ha portato il maggiore partito della maggioranza dalle posizioni iniziali fino alle posizioni di fine legislatura. Vi invito a ricordare ciò che è accaduto all'inizio

Partito Democratico pensò di poter passare in forza, dopo aver rottamato la sinistra *post* comunista e filo CGIL, e di poter trasformare il nostro sistema istituzionale istituzionale riducendo ad una le Camere del Parlamento e varando una legge elettorale che prevedeva l'elezione al secondo turno del Presidente del Consiglio e, caso unico nella storia - come dissi a Renzi in una riunione in una riunione del PD - questa elezione nel doppio turno del candidato Presidente, gli dava automaticamente diritto ad un premio di 140 deputati nell'unica Camera. Da questo punto di vista, se tale sistema se tale sistema di riforme costituzionali fosse passato, avremmo avuto il tipo di governabilità che poco fa il presidente Napolitano riteneva e definiva scompensata e non equilibrata,

Mettiamola così. Sappiamo che la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l'Italicum proprio in quel punto, nel doppio turno con l'elezione del Presidente del Consiglio diretta, come sottolineato anche dal

allontanato momentaneamente da Palazzo Chigi, per tenere caldo il posto e che invece si è accreditato, guadagnandosi l'appoggio del Presidente della Repubblica, la stima

italiana. Quando dissi a Renzi che nessun Paese di democrazia occidentale aveva una legge come l'Italicum e che quindi si sbagliavano i professori che lo avevano consigliato - Ceccanti e D'Alimonte - egli capì subito al volo e disse: non ce l'ha nessun altro Paese, ma tutti ce la imiteranno. Non è così: non si possono distruggere i sistemi istituzionali *ad libitum*. Da questo tipo di narrazione, si è passati infine ad un'altra, ovvero al ritorno di Ghino di Tacco. Il problema fondamentale della prossima legislatura sarà infatti quello di avere un gruppo di fedelissimi, con cui "vendere cara la pelle", porre il dazio a tutti gli altri, essere l'elemento che non può governare, ma che impedisce ad altri di governare e che quindi ha un potere di interdizione molto forte. Come hanno detto molti colleghi, è possibile che la Corte costituzionale dichiari illegittima

in condizioni particolari, dopo una battaglia durissima, un'altra cosa è la fiducia preventiva, generalizzata, che impedisca in assoluto l'emendabilità di tale legge. In tal caso c'è un potere democratico, quello del Governo, che prevarica un altro potere, quello del Parlamento. Anche in

ingovernabile e ancora una volta delegittimato. Condivido le preoccupazioni di chi dice che continuare con questo spirito antiparlamentare arreca un danno all'Italia, perché non c'è un'alternativa. Nei momenti rivoluzionari si

Mi rivolgo ai colleghi del Gruppo Partito Democratico, con cui fui eletto ormai quasi cinque anni fa e con cui ho lavorato, costruendo spesso rapporti di stima e di amicizia personale, dicendo

Trovo un po' vigliacco parlare del peccato e non del peccatore. *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Chi sta facendo pressione sul Presidente del Consiglio? Sarebbe il caso in un momento così delicato della vita democratica di questo Paese avere una visione

perché, in fondo, il Partito Democratico ha paura dei franchi tiratori. Poi Forza Italia esce, la Lega si defila e noi consegniamo al Paese una legge elettorale che vogliono tutti, ma che non riconosce nessuno. Io lo trovo veramente poco onorevole, anche a discapito di chi la dovrà in qualche maniera giustificare. Posso capire la Lega la Lega che ha fatto il suo "accordicchio" per prendersi quattro seggi in più nel Nord Italia e se ne va a casa contenta, nonostante abbia tradito completamente qualunque forma di

Forza Italia, Lega e Movimento 5 Stelle. Allora, Lega e Forza Italia, che non vanno d'accordo apparentemente su nulla, sono disponibili. Ciò lo dico anche al collega Orellana,

vogliono coloro che andranno a votare nel momento in cui avranno capitalizzato il "voticchio" del cacciatore, dell'animalista, del pensionato e dell'imprenditore tutti insieme. Da una parte la Lega dice di voler eliminare la legge Fornero sul pensionamento

tutti immobili e fermi assistendo alla distruzione del Paese Italia e noi siamo costretti per la disperazione a compiere azioni di cui non andiamo fieri. A me non me ne frega niente di sedermi lì e bloccarvi i lavori,

che stanno cercando di dire che non sono né ciechi, né muti, né sordi. È così che ci volete, ma qui dentro non c'è peggior sordo di chi non vuol sentire.

Signor Presidente, il Gruppo di Forza Italia, com'è noto, è favorevole a questa legge elettorale. I Regolamenti di Camera e Senato sono diversi, quindi il voto di fiducia, che qui assorbe anche quello nel merito sull'articolo,

come i colleghi sanno, il voto di fiducia poi viene seguito da quello di merito - abbiamo potuto differenziare il nostro atteggiamento. La situazione quindi è molto chiara per noi: no alla fiducia, condivisione della legge. Ci regoleremo come le norme del Regolamento ci consentono di fare, senza alimentare, con voti di fiducia inutili o impropri, una situazione di confusione, perché poi l'elettorato deve capire che un conto sono le regole e un conto è il merito politico.

di merito, sul voto disgiunto o no. Le abbiamo sperimentate tutte le leggi elettorali, perché anche all'epoca del Mattarellum, che era simile a questa (anche se il dosaggio dei due terzi e di un terzo era l'inverso,

vero, senza recupero proporzionale, senza niente. Alla fine, perfino il sistema inglese si è logorato e non so nemmeno che fine abbiano fatto i conservatori che hanno vinto: li abbiamo lasciati che inseguivano alcuni eletti irlandesi - o gallesi, non lo ricordo esattamente - per avere la maggioranza in una delle

allo stato, il centrodestra potrebbe avere anche la maggioranza assoluta dei consensi. Lo scopriremo quando si voterà e nessuno deve immaginare che la legge elettorale sia fatta a proprio modello. Chi lo ha fatto - e tutti lo abbiamo fatto a fasi alterne - poi si è trovato a fare una legge elettorale che ha fatto vincere gli avversari. Ma questo è il bello della democrazia: la non

storia del mondo e le cose devono essere tutte studiate e discusse. Francamente ho trovato un po' strano che si sia fatto un microdibattito e ringrazio il senatore Mario Mauro, che ha preso la parola per ripristinare alcuni fatti di verità. Ora il senatore Tronti, che ha seguito i lavori della mattina,

Quindi potrebbe essere - con una battuta - cugino di Pol Pot? Credo di no, perché tra Pol Pot e Tronti la differenza mi è assolutamente evidente, non voglio quindi accomunarlo. Ma dico al professor Tronti che tutti i totalitarismi devono essere messi al bando. Oggi noi non faremmo la discussione sulla legge elettorale - bella o brutta, cari colleghi, ma è una legge elettorale, la gente voterà - se avessero vinto i totalitarismi del secolo scorso, tutti i totalitarismi. Stiamo parlando in ore in cui giustamente tutta l'Italia condanna alcune forme becere e intollerabili di propaganda nazista, ma varrebbe lo stesso se parlassimo di altri totalitarismi. Alcuni hanno chiamato la legge il «fascistellum», anzi, hanno detto che era quasi più democratico il modo di votare prima. Tutti i totalitarismi devono essere messi al bando, di ogni colore e orientamento. Non parlo, quindi, in nome di una parte, ma francamente consiglio al professor Tronti di rileggersi l'edizione originale de «Le livre noir du communisme», il libro nero del comunismo, che uscì in Francia - questa è l'edizione autentica, poi fu ristampato

di cui proprio in queste ore si sta parlando, ricordando lo sterminio, l'Olocausto e quant'altro, per le vicende sciagurate che si sono verificate, anche quella rivoluzione di cui Tronti si sente figlio oggi non ci avrebbe consentito di fare una discussione sulla legge elettorale, perché non ci sarebbe stata la possibilità elettorale. Anche con altri totalitarismi sarebbe stata la stessa cosa.

approvata. Francamente ho trovato discutibile questa rievocazione, anche quando si diceva che è stata fatta in omaggio ad alcuni Padri costituenti. Non voglio aprire a quest'ora, in una giornata particolare, il dibattito su Togliatti, che è stato in Russia mentre gli italiani venivano uccisi; anche qualche Padre della Patria è stato patrigno della Patria in alcuni momenti. Vorrei che restasse agli atti che è giusto ricordare e discutere la storia, ma che quella storia, se fosse stata vincente, non avrebbe portato democrazia, come altre storie: i milioni di morti, i massacri che si sono verificati non devono essere dimenticati. Quindi, contento contento il senatore Tronti di essere figlio di quella storia, contento io che oggi ci sia un libero Parlamento in cui ciascuno può dissentire, anche facendo le manifestazioni fuori, se avvengono pacificamente. Per la verità ce ne sono state alcune, signor Presidente, un po' antipatiche, perché non è bello, colleghi, mettere le foto delle persone e indicarle, come ha fatto qualche collega anche del vostro Gruppo. con riti: si parla della Rivoluzione di ottobre, salto a quella successiva, quella maoista. Ci può essere la polemica o la manifestazione, ci mancherebbe altro; chi di noi non ha dissentito, ma *est modus in rebus*. Mi auguro, allora, che il senatore Tronti abbia il tempo di rileggere qualche libro importante e di dire che forse è meglio essere figli della democrazia e non della Rivoluzione d'ottobre.

una rappresentante del Movimento 5 Stelle, credo dopo aver esaurito una serie di più significative curiosità, pensato di chiedermi pubblicamente come la pensassi a proposito della grave questione che stiamo dibattendo. Prenderei le mosse dall'intervento di ieri del collega illustre

con l'intenzione di collegare fenomeni, eventi, esperienze lontane a qualcosa che ha la qualità per resistere alle cose che noi stiamo dibattendo in questi giorni, per la verità con la difficoltà di trovare una sorta di memoria dei modi di rappresentare le idee,

del nostro illustre collega di risvegliare qualcosa di sé stesso, che in una certa misura ritrova vaghe assonanze nelle questioni sulle quali ci troviamo impelagati da qualche tempo. Mi riferisco all'*incipit* apparentemente inopinato di un intervento che partiva dalle ragioni della sua antica passione politica e ideale. È per lo stesso motivo che oggi, convertito dalla contemporaneità

a manifestare le sue idee sulla politica in una maniera non distante, né rinnegatoria, di cose vissute nella sua vita più giovane,

colma di una sorta - passatemi l'espressione - di redenzione razionale che lo accompagnasse nel seguito di una laboriosa attitudine al rispetto dell'errore,

se non per riconoscere che l'idea dell'errore, nella nostra fugace storia quotidiana, deve indurci a conservare quella ricchezza generale che è il dubbio, cioè l'intelligenza del confronto, del contrasto, della distinzione, i tre segni del procedere critico del pensiero, a garanzia che non prevalgano le ragioni solo oppositive. E qui mi tengo alla coraggiosa e penetrante saggezza di Giorgio Napolitano. Il suo a ritrovare il valore indicibile della comunità, con le riserve democratiche, insieme, della condivisione e dell'opposizione.

alle premesse e allo stigma della libertà. Ho improvvisato qualche appunto, perché mi sono sentito in obbligo di dare una risposta alla collega

anziché dedicarvi l'attenzione, l'impegno e la tensione anche morale ed etica che meriterebbero, trattandosi di problemi come quelli che abbiamo trattato fino a oggi, quasi non fossimo più tenuti a rispettare la necessità la necessità di vivere con gli altri, di rappresentare una civiltà che si muove, si giustifica e cresce soltanto in funzione di viverla insieme. Don Milani disse che «la politica è uscirne insieme»: non voleva dire una cosa generica o soltanto virtuosa voleva dire semplicemente che ciascuno di noi da sé è la metà di ciò che dovrebbe, che l'altra metà è l'altro. Quando mi fu chiesto - scusate se mi intrattengo su un particolare personale che non ha alcun rilievo per le vostre conoscenze,

dal mettersi insieme a rivedere cose, a giudicarle e a tentare di trovare un vicolo che attraversi - perché no?

dell'argomento, delle sue articolazioni anche di carattere storico perché ha voluto richiamarsi a esperienze passate.

ha prodotto, vi è tuttavia qualcosa che contribuisce a fornirci gli elementi per rivedere le nostre persuasioni;

Credo invece che sia una buona ragione quella un po' pedissequa, o forse banalizzante, del non prendere sul serio tutte le cose, anche quelle che ci paiono solo strumentali.

ci paiono solo strumentali. Spero che questa circostanza servirà a ricreare un clima che deve corrispondere alla serietà e alla dignità di questo luogo,

credo di soffrirne come tutti voi. Ho grande stima e rispetto per il valore indicibile della costanza e della pazienza che manifesta il Presidente del Senato mi chiedo se non vi sia un motivo molto serio per rivedere, anche in nome della serietà personale di ciascuno di noi, le questioni che ci tengono lontani, come se fossimo qui a fare una guerra, anziché cercare una pace sociale, civile, culturale. Tanto che Giorello,

Credo che, se decideremo di far parte di un mondo che si salva soltanto mettendosi insieme e unendo le forze, si possa

Abbiamo ancora il tempo per mettere a posto le cose e non dovremo credere che, risolta con il voto di fiducia tale questione, essa perciò stesso sia risolta. La questione rimane in piedi, con tutto il carico del tempo perduto, delle offese gratuite e del bisogno qua e là di cercare gli spazi del populismo che hanno

alla Camera qualche mese fa, non noi ma altri, hanno scelto di far saltare una legge elettorale disegnata sul modello tedesco. Su quella legge vi era un ampio accordo.

Le ragioni cui il Presidente della Repubblica ci ha spesso richiamato restano tutte in campo. C'era e c'è la necessità di una legge elettorale che omogeneizzi i sistemi di Camera e Senato per ridurre l'ingovernabilità. C'era e c'è la necessità di una legge che restituisca forza alla rappresentanza di genere. C'era e c'è la necessità di una legge elettorale fatta dal Parlamento e non di risulta sulle sentenze della Corte costituzionale.

mesi ci hanno accusato di non voler fare la legge per favorire l'ingovernabilità e l'inciucio. Oggi gli stessi ci accusano di aver fatto una legge elettorale per favorire l'inciucio. In realtà, non abbiamo mai smesso di lavorare per rispondere ai richiami giusti del Capo dello Stato, guardando all'interesse del Paese. Oggi ci troviamo in Aula con un disegno di legge approvato alla Camera dei deputati con - lo voglio sottolineare a chi ci dà lezioni di democrazia

serviva e serve una legge elettorale in cui gli elettori possano scegliere chi governa e che garantisca a chi è

oggi, che introduce una quota di maggioritario importante, favorendo l'aggregazione di forze che condividono proposte e progetti per il futuro e riducendo i rischi di ingovernabilità. Questa è una legge che, allo stesso tempo, garantisce la rappresentanza di genere e, comunque, la rappresentanza dei territori. È una legge costruita

A chi grida allo scandalo, teorizzando che solo le preferenze consentono la scelta ai cittadini, voglio ricordare, innanzi tutto, che l'accordo che avevamo fatto tutti sul sistema tedesco prevedeva i capilista bloccati. in una parte del Paese, le preferenze possono consentire, come abbiamo troppo spesso visto, condizionamenti che con la libertà di scelta e la libertà degli elettori hanno poco a che fare. Questo è a che fare. Questo è il momento, come richiamava anche il presidente Napolitano, della responsabilità. Non è il momento della propaganda, in cui, dopo aver criminalizzato il voto segreto, oggi si teorizza che esso dovrebbe diventare la regola e se ne propongono quarantotto. Serve una legge elettorale nuova, fatta dal Parlamento. Tra poco sarà sconfitto chi, invece, una legge non la vuole, come ha dimostrato affossando il sistema tedesco e dicendo tutto e il suo contrario, pur di lasciare le cose come stanno. Ripeto, questa è la miglior legge possibile in questo Parlamento. Per farla, ognuno dei suoi sostenitori, ognuno di coloro che la voterà ha rinunciato a qualcosa. Tutti insieme, però, una larga maggioranza di questo Parlamento, abbiamo fatto prevalere e faremo prevalere l'interesse del Paese. del Paese. Come chiedeva il Capogruppo del Movimento 5 Stelle ci sarà traccia di questa discussione. Ci sarà traccia e sarà quella lasciata da una maggioranza e da una grande parte dell'opposizione che, come si deve fare sulle regole, hanno condiviso questa legge elettorale e si sono assunti la responsabilità di farla.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

Mauro Maria,

Prego di evitare le provocazioni e le reazioni.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

Contrari | 61 | **Il Senato approva.** Risultano pertanto preclusi tutti gli emendamenti e gli ordini del giorno presentati all'articolo 3 del disegno di legge n. 2941. Passiamo ora alla votazione dell'articolo 4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

Presidente, io non so cosa stiamo votando; non so se stiamo votando le coperture finanziarie o una copertura delle vergogne. La nuova ammucchiata del Governo Renzi-Verdini-Alfano - abbiamo visto passare oggi la nuova maggioranza - con l'assistenza complice di Salvini e Berlusconi, con l'apposizione

Hanno lasciato questo articolo come una microscopica aiuola, un albero stentato nel parcheggio di un ipermercato delle vacche. Per chiedere tutte queste fiducie bisogna essere credibili. «È la prima volta che mi capita di non dare la fiducia ad una persona come te, ma non perché sei tu, ma per quello che rappresenti. Tu rappresenti le banche, i poteri forti, dici una cosa e la smentisci il giorno dopo. Sei un ragazzo giovane ma allo stesso tempo vecchio, noi siamo l'opposto». Ve le ricordate queste parole? Sono quelle che Beppe Grillo ha pronunciato in faccia al presidente eletto da nessuno Matteo Renzi. *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Voi, invece, avete continuato a dargli fiducia quando ha umiliato la scuola, devastato il mare con le trivelle petrolifere, precarizzato e soggiogato i lavoratori, abbandonato i risparmiatori truffati proprio dalle banche. Il 4 dicembre scorso i cittadini l'hanno mandato a casa per aver tentato di distruggere la nostra Costituzione. Voi avete dato continuità al suo progetto scellerato e ora votate la fiducia su un disegno di legge elettorale che vi condanna agli occhi degli italiani e di tutto il mondo civilizzato. Dovevate mettere la fiducia su tutto il disegno di legge. E invece no, perché altrimenti sarebbe tornato alla Camera dei deputati e avete paura delle elezioni in Sicilia. A voi dico che a votare sui vostri specchietti per le allodole non ci stiamo. Il Movimento 5 Stelle lascerà quest'Aula in questo momento. siciliani dico che il loro voto può cambiare il corso delle cose non solo per la loro Regione, ma per salvare l'Italia intera. So che molti di voi sono al Pantheon. Vi raggiungo là e parleremo liberamente. Le istituzioni siete voi.

«Diciamo che manterremo il figlio passandogli l'assegno mensile. Non vogliamo che muoia fino alla scadenza naturale».

Romani. Qualcuno gli chiede: perché lei e Zanda siete inseparabili? «Ci sentiamo molte volte al giorno, anche la domenica». Questa legge, dopo aver letto questa sceneggiatura, è il frutto - e non c'è niente da ridere - dell'orgia Verdini-Renzi-Berlusconi, con Zanda maggiordomo a reggere la candela e Alfano a fare il palo dietro la porta! Tutto il sistema si è attivato per proteggere la propria poltrona e il vitalizio. Tagliatevi i vitalizi e non la democrazia! Questo è ciò che dovreste fare. Infine, presidente Grasso, l'appello glielo abbiamo rivolto in molti. Nel lontano 1953 il presidente Paratore, davanti alla richiesta di fiducia - dopo averla suo malgrado concessa, perché non poteva fare altrimenti - prima che venisse votata, si dimise e fu il Vice Presidente a porla in votazione. È l'ultima occasione, l'ultima speranza, l'ultima possibilità per fermare questi abusivi del Parlamento. Signor Presidente, non si renda complice. *(Applausi

non ho bisogno di medaglie ma ho il senso delle istituzioni. Come tutti sanno, il motivo per cui non ho accettato la candidatura in Sicilia è stato per potere continuare, con senso delle istituzioni,

a larghissima maggioranza. Pensavamo, quindi, che quel voto avesse ridato forza non solo al Senato ma alla nostra Costituzione e siamo arrivati a questa discussione - prima ancora in Commissione - con

- è successo tante volte in questa legislatura - ci siamo trovati di fronte a un voto di fiducia. Per la verità, non ci saremmo mai aspettati che sulla legge elettorale si ponessero tre fiducie alla Camera e cinque al Senato.

Tutto questo non solo non fa bene a questa istituzione, non fa bene alle istituzioni democratiche, Presidente. Non farà bene alla politica italiana, perché ancora una volta i cittadini fuori da

un sistema di potere, un sistema politico che, ancora una volta, com'è successo con il *referendum*, sarà smentito dalle elezioni. Abbiamo visto che le quattro fiducie

Signor Presidente, oggi abbiamo assistito ad una prova di forza. Il cartello - perché di questo si tratta - che ha sostenuto la legge elettorale, l'ha imposta al Parlamento e in particolare al Senato, senza alcuna possibilità di confronto e di dibattito, con il ripetersi di voti di fiducia,

dal senatore Verdini, noto come ALA, è entrato a far parte della maggioranza, votando ripetutamente la fiducia, nonostante questo aiuto la maggioranza che sostiene il Governo non è una maggioranza assoluta.

come ci raccontava questa mattina il presidente emerito Napolitano, costretto dalle pressioni di una qualche maggioranza non ben identificata. Un Presidente del Consiglio, infatti, non prende nessuna decisione costretto da altri, ma si assume da solo

Quindi, il Governo, capeggiato dal presidente del Consiglio Gentiloni Silveri, ha scientemente deciso di esporsi in quest'Aula allo scempio di cinque voti di fiducia sulla legge elettorale, rispetto alla quale, com'è stato ripetuto a iosa nel dibattito che ha preceduto questa votazione, aveva sempre detto che si sarebbe tenuto perché trattasi di legge squisitamente parlamentare. Si è quindi preso il rischio di essere nella situazione in cui si trova ora: una situazione in cui ha registrato che la sua maggioranza è una minoranza e che, da ora in poi, a partire dal delicatissimo passaggio della legge di di bilancio, se vorrà avere una maggioranza, dovrà pietire il sostegno - fatto, come oggi si è visto, di missioni finte, di malattie impreviste e presenze non dichiarate - di un'altra forza importante: Forza Italia. Non è un caso che sia avvenuto ciò e quanto è accaduto oggi in Assemblea lo rende palese. La nuova maggioranza che si è andata costituendo, una maggiore silenziosa, che non si appalesa nel voto di fiducia,

Abbiamo provato con le armi di cui disponiamo. Abbiamo votato convintamente no su tutti gli articoli che evidenziano le distorsioni e le assurdità di questa legge elettorale.

Presidente, abbiamo parlato finché c'era qualcosa da dire e abbiamo ascoltato finché c'era qualcosa da ascoltare. Ora, come ho annunciato

della nuova maggioranza di Governo che abbiamo visto affiorare ogni tanto dalla melma che la nascondeva e quelle di chi in coscienza, nei corridoi, ha avuto il coraggio di ammettere con noi che questa legge è inaccettabile. Vedremo qui che cosa faranno, ma lo vedremo dopo. Noi adesso andiamo in piazza con i cittadini. RUSSO *(PD).* Non

La *ratio* di questa norma è che i cittadini italiani che vivono in quelle terre vengano eletti in queste sterminate circoscrizioni estere per portare nel Parlamento italiano la voce dei nostri migranti. Può essere una scelta giusta o sbagliata, ma abbiamo costruito queste circoscrizioni, che non costano poco, perché è evidente che organizzare le elezioni nella Terra del fuoco in Argentina, negli Stati Uniti o in Canada, in Australia, in Europa o in Africa, ha un costo. La Camera ha deciso

e aver stabilito che i rappresentanti dei nostri migranti devono venire qui a dare voce a chi vive lontano, ma si sente italiano, adesso invece stabiliamo che nelle circoscrizioni estere va a fare campagna elettorale chi ha sempre vissuto in Italia ed è residente nel

che è successo

La seduta è tolta